*(PD)*. Signor Presidente, le ho chiesto la parola in apertura di seduta

Il tema è quello riguardante la sorte di persone inermi, costrette su una nave, la Sea-Watch 3, a poche decine di metri dal porto di Siracusa nel mare italiano e in territorio italiano. È una sorte che porta la gran parte degli italiani ad un'indignazione per l'insopportabilità di vedere impedito dalle autorità del Governo italiano lo sbarco e l'attracco della Sea-Watch, a bordo

di chi fugge da guerre e da maltrattamenti indicibili. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Signor Presidente, noi parlamentari del Partito Democratico ieri eravamo nel porto di Siracusa. Tra quei parlamentari c'erano i senatori del Partito Democratico - oltre al sottoscritto, il senatore Davide Faraone e la senatrice Valeria Sudano - per chiedere

la dignità del nostro Paese che in questi anni ha salvato migliaia di vite nel Mediterraneo, riscattando anche la coscienza europea

Sono saliti a bordo di quella nave i due capi della nostra delegazione, il presidente del Partito democratico Matteo Orfini e il deputato Maurizio Martina. Hanno potuto verificare le condizioni insostenibili, non sono delle 47 persone, soprattutto dei minori, ma anche dei 22 membri dell'equipaggio; insostenibili per motivi igienici, sanitari ed anche psicologici. Una volta tornati a bordo, sia l'onorevole Orfini sia l'onorevole Martina hanno saputo di essere indagati. Ecco noi, Presidente, siamo molto colpiti da questo, ma non siamo turbati. Noi abbiamo fatto e faremo valere le prerogative dei parlamentari *(Applausi dal Gruppo ma il dovere di intervenire a nome di tutto il popolo italiano in questi casi e sempre. Non siamo turbati anche, signor Presidente, perché la visita a bordo della Sea-Watch 3 che abbiamo effettuato ha seguito un incontro che, come delegazione dei parlamentari del noi, signor Presidente, abbiamo avuto con il prefetto e alla presenza del prefetto con il comandante della Capitaneria del Porto di Siracusa, che è la massima autorità marittima. Abbiamo concordato alla presenza del prefetto, con la massima autorità marittima, di visitare la nave, affittando un natante privato *in* *loco* dal porto di Santa Panagia. Abbiamo svolto la nostra visita con estrema correttezza il rispetto di tutte le regole. Per questo, Presidente, non siamo turbati, ma siamo assolutamente indignati invece per l'atteggiamento del Governo italiano. Riteniamo che questo atteggiamento stia violando e calpestando le leggi dello Stato italiano che dicono che di fronte a dei minori non accompagnati non ci può essere alcun respingimento. Nessun minore può essere tenuto al largo al rischio della propria vita. Non siamo turbati e per questo, Presidente, depositeremo in questi minuti un esposto alla procura di Siracusa contro il Governo italiano per violazione delle leggi italiane *(Applausi dal Gruppo PD)*e del nostro Stato di diritto. Presidente, colleghi, non c'è alcuna sicurezza per gli italiani lasciando morire in mare persone inermi. Non risolveremo alcuno dei nostri problemi lasciando al largo persone che hanno il diritto di sbarcare e soprattutto non cambieremo l'Europa isolandoci. Vogliamo cambiare l'Europa; vogliamo che l'Europa si occupi ed abbia una politica unica sull'immigrazione. Lo abbiamo voluto e fatto durante i nostri Governi. Vogliamo che avvenga anche con questi Governi. Per questo noi eravamo a Siracusa ieri e saremo a Siracusa oggi. I parlamentari del PD continueranno ad essere a Siracusa finché non scenderanno tutte le 47 persone a bordo, finché non scenderanno quei minori, affinché non accada più la vergogna che sta accadendo in queste ore, per riscattare l'Europa e l'Italia che sono grandi potenze economiche perché, signor Presidente, sono innanzitutto grandi potenze morali. Questo fa grande la nostra politica, la nostra economia e il nostro *made in Italy*: la possibilità per il popolo italiano di potersi riconoscere in un Governo

ma, signor Presidente, non deve appartenere a nessuno in quest'Aula, perché non appartiene a nessuno nel popolo e tra i cittadini italiani.

dopo l'iniziativa dei tre parlamentari (il mio segretario e i deputati Maggi e Prestigiacomo),

Ancora una volta ci troviamo di fronte a una situazione incredibile, un copione che ormai si ripete continuamente. Mi riferisco al fatto che, da parte del Governo italiano, non c'è alcun tipo non

che ci nega perfino l'ospitalità della sabbia; che ci dichiara guerra e ci vieta di posarci sulla vicina terra. Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia mortali, credete almeno negli Dei, memori del giusto e dell'ingiusto». Queste parole

di uomini è mai questa?». Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia mortali, credete almeno in Dio, memore del giusto e dell'ingiusto.

E questo noi continueremo a fare, con atti come quello che ha compiuto il segretario del mio partito Fratoianni, insieme ad altri parlamentari, non per fare testimonianza, ma per denunciare e svolgere fino in fondo le nostre prerogative di parlamentari, perché noi innanzitutto non dimentichiamo di essere umani. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, anche noi abbiamo un cuore e non pensiate che non ci sia sofferenza nel vedere queste situazioni drammatiche che si verificano ai confini della nostra nazione (figuriamoci). Siamo un partito che ha fatto della libertà e dell'umanità una bandiera sempre innalzata. Ma oggi dobbiamo fare i conti con un problema diverso: il problema

Noi abbiamo sempre avuto, signor Presidente, una posizione di grande equilibrio e abbiamo al contempo un'idea forte che ci conduce, quella di mantenere la sicurezza all'interno del nostro Paese. Abbiamo fatto grandi sacrifici come popolo italiano e ci dispiace quando sentiamo qualcuno che ci definisce razzisti o che dice addirittura che non stiamo facendo il nostro dovere come popolo italiano. *(Applausi dal Lo stiamo facendo con le nostre tasse e con il nostro aiuto; abbiamo avuto un approccio di accoglienza che nessun altro Paese europeo ha avuto. Ed è per questo che io credo che noi dobbiamo a questo punto valutare politicamente quanto si è verificato. Abbiamo chiesto aiuto all'Europa e l'Europa cosa ci ha risposto? Ha chiuso i confini. Lo hanno fatto l'Austria e la Francia (ce li rimandano addirittura indietro); e potrei continuare. Dov'è questa solidarietà che l'Europa sbandiera e che poi ci nega, che nega a un Paese importante come l'Italia? Noi stiamo gestendo da anni questo dramma e lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Voglio ricordare e ringraziare soprattutto il nostro presidente Tajani per le politiche che ha applicato. Il Presidente del Parlamento europeo ha votato - lo voglio ribadire e sottolineare - la modifica al Trattato di Dublino. Ma dov'era il Consiglio d'Europa? Dov'era la Commissione europea? Perché non è stato fatto un passo analogo a quello fatto dal presidente Tajani? Sono queste le ragioni per le quali io credo

attuare una politica certamente di apertura per quanto abbiamo fatto qui in Italia, ma soprattutto di grande consapevolezza di quella che è la realtà. Un segnale di apertura in quelle terre porterebbe ancora a nuove partenze; e nuove partenze significherebbero nuovi morti. Noi, quindi, alla politica delle porte chiuse dell'Europa non possiamo rispondere con la politica delle porte aperte dell'Italia.

parere della 5a Commissione. Invito i relatori a prepararsi sui pareri, in modo che vengano espressi in maniera rapida e precisa. *(La seduta, sospesa

trovammo un emendamento pericoloso, con una parte che procurava alle casse dello Stato 120 milioni di euro: era la parte che raddoppiava

ma la cultura e il significato politico che da sempre il volontariato ha avuto nel nostro Paese. C'è qualcosa di buono che resiste al passaggio e al trasformarsi della società ed è proprio il forte radicamento di questa passione per gli altri: il Governo, però, con una parte della legge di bilancio ha deciso, in maniera inconsulta evidentemente, di penalizzarlo con violenza di umiliarlo di fronte all'opinione pubblica, raddoppiando le imposte a tutto il mondo *no profit*. Non si può dire che non lo sapevano e che non si stavano rendendo conto di quello che facevano, perché abbiamo avuto modo di

ha deciso di raddoppiare le tasse sulla bontà, quasi che la bontà fosse un lusso, una cosa pericolosa, perniciosa per il futuro del nostro Paese. Queste sono le scelte che avete fatto. Poi, finalmente, è tornato il buonsenso, forse per la reprimenda del Quirinale, forse per la rivoluzione che si è creata nel Paese sulla vicenda; forse per lo scandalo che il Partito Democratico ha voluto denunciare con forza nelle settimane successive all'approvazione. PD)*. Sono disponibile a riconoscere ai Presidenti dei Gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega di aver collaborato in questa fase di esame del provvedimento e di aver fatto in modo di trovare i fondi per sanare quella ferita gravissima che avete inferto al nostro Paese; quella ferita vergognosa che, in occasione della legge di bilancio, la legge più importante di politica finanziaria varata nel nostro Paese, avete voluto infliggere.

emendamenti intervenuti per sanare la vicenda - è una proposta sacrosanta, forse la parte nobile di tutto questo provvedimento vergognoso e affazzonato che ci permette di guardare in faccia

del Parlamento contro la volontà negativa che il Governo ha dimostrato nella legge di bilancio. Signor Presidente, colleghi tutti, vi ringrazio per la disponibilità rispetto al voto favorevole a questo emendamento. Credo che finalmente il Parlamento abbia riacquisito

si riacquisti finalmente la dignità del Senato della Repubblica, la dignità del Parlamento tutto, e si riprenda a lavorare nell'interesse della nostra comunità nazionale.

bisogna evitare la superficialità, soprattutto quando si parla di questioni così fondamentali. Se invece - lo dico per ciò che potrà succedere il prossimo anno - ci fosse la volontà di mettere in discussione questa

durante la quale i nostri emendamenti sono stati puntualmente respinti. Su questo tema vi è stata una convergenza nelle Commissioni riunite a seguito della presentazione di identici emendamenti da parte di tutti i Gruppi; ragion per cui non abbiamo avuto

i docenti del Liceo classico «Gabriele D'Annunzio» di Pescara, che stanno assistendo ai nostri lavori dalla

Pur mantenendo tutti i requisiti previsti dalle SOA, abbiamo chiesto un periodo di transizione, concordato per un massimo di dodici mesi, per garantire a quelle aziende di poter partecipare alle gare d'appalto. Tengo a sottolineare il fatto

e con l'emendamento 1.0.21, dichiarato ammissibile. Apprendiamo poi che la maggioranza lo accoglie e lo copia con un proprio emendamento; ne prendiamo atto con piacere, ma Fratelli d'Italia rivendica

G3.79 è accolto come raccomandazione, a condizione che si riformuli espungendo il punto 5. Esprimo

perché si pone in continuità con le scelte che abbiamo portato avanti nella passata e nell'attuale legislatura per garantire trasparenza, tracciabilità e certezza ai consumatori il contenuto dei prodotti che vengono messi loro dinanzi. Voteremo favorevolmente perché il decreto che dovrà essere emanato sarà sottoposto al vaglio

dichiarazione di voto anche per esprimere soddisfazione per il fatto che sia stato ritirato l'emendamento 3.0.500, che rimetteva in discussione il bando SIAN, perché ci ha evitato di fare una scelta che avrebbe potuto comportare conseguenze molto pesanti al settore agricolo, sia per i rischi di illegittimità che comportava quel tipo di provvedimento, sia per tutti gli interessi che andava a rimettere in gioco. Non sto qui a soffermarmi su tutto quanto hanno espresso nei giorni scorsi i giornali specializzati in materia. Credo che revocare una gara da oltre 300 milioni di euro, dichiarando, nella relazione che c'era stata data al Senato, che la verifica non era conclusa, quando a ottobre del 2018 la Consip, incaricata dall'Agenzia confermava il soggetto vincitore, che, avendo vinto, aveva verificato i requisiti sia di competenza che finanziari e li trovava a posto, sia stata una forzatura e una disinformazione, fatta a questa Assemblea, che, a parte coloro che si sono occupati specificatamente della materia, sarebbe sfuggita. Credo che, anche da parte degli Uffici del Senato, simili scivolate non dovrebbero più succedere. Abbiamo rischiato di invalidare un bando di gara sulla base di errate informazioni, che non ci hanno messo nelle condizioni di votare consapevolmente. Poi, per fortuna, ieri è intervenuto il ritiro di quell'emendamento e abbiamo scampato il pericolo.

una decina di anni di lavoro e di tentativi. Ricordo nel 2010 un disegno di legge della Lega sull'etichettatura e poi, dopo ben cinque Governi targati PD, oggi il Governo

tutti quanti noi. Dopo dieci anni, finalmente, avremo un po' di trasparenza sulle tavole di tutti i cittadini del Paese e avremo dato un po' di verità sulle etichette dei nostri prodotti agroalimentari.

anche per le imprese balneari, che sono un pezzo dell'economia produttiva, del turismo, della vivibilità e della qualità del nostro territorio, ferme restando corrette regole di utilizzazione delle spiagge? Riteniamo che la vicenda non sia finita e che si debba arrivare alla loro totale esclusione. Nel frattempo, in esame, sopravvissuto alla selezione sul campo a differenza di altri, chiediamo un segnale a favore di tale settore, per il quale continua l'impegno di Forza Italia per giungere alla sua esclusione totale dalla direttiva Bolkestein, così come si è verificato per il commercio ambulante. Siamo lieti per loro, ma non vogliamo che sia penalizzato un altro settore produttivo importante. Quest'emendamento è un segnale sul tema: chi vuole difendere il mondo balneare, lo approvi; chi è contro, lo bocci. Non si sfugge.

e lo sta continuando a fare. Dobbiamo però soffermarci e cercare di comprendere meglio le regole per tenere dentro tutti, ma per farlo nella maniera migliore ce ne occuperemo nei prossimi giorni, magari con un decreto *ad hoc*.

l'emendamento 3.0.81. A me non risulta che da parte delle categorie economiche ci sia stata la richiesta di allungare i termini per evitare un reato penale, portandoli da tre mesi, successivi all'accertamento

Signor Presidente, cari colleghi, mi permetto di rinnovare il mio appello, già avanzato in Commissione,

prestazioni di lavoro occasionale per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali. La medesima disciplina è già prevista per le società sportive che possono far uso dei *voucher* per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. Allora, perché - mi chiedo e ci chiediamo come Gruppo per le Autonomie - non estendere tale disciplina anche agli enti *no profit* che perseguono le stesse finalità? La materia del lavoro in generale e la materia del lavoro occasionale, in particolare, non è il dominio di un partito o in particolare di un movimento politico. Perché, quindi, non valutare proposte che, come questa, sono di buon senso? Faccio l'esempio più noto, al quale se ne potrebbero aggiungere molti altri: nel 2020 ci saranno le Olimpiadi invernali e alcune di queste gare - le gare di biathlon - si svolgeranno ad Anterselva. L'organizzazione delle gare ad Anterselva è in capo al biathlon Anterselva, vale a dire un'associazione *no profit* che non è in grado di organizzare l'evento

ad organizzare meglio eventi e manifestazioni sportive di una certa rilevanza, potendo usufruire, per periodi anche brevi, di strumenti come i *voucher* per far fronte

in tema di modi della custodia. Al settimo comma dell'emendamento si dice che «Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione». Vorremmo conoscere dalla relatrice, ed eventualmente anche dal Governo, il motivo

dell'immobile, il divieto di dare in locazione l'immobile stesso è lasciato solo per il debitore, ovvero si prescrive che il debitore possa concedere in locazione solo se autorizzato dal giudice.

Presidente, parliamo di semplificazione. Credo che l'osservazione fatta dal collega Cucca sia di buon senso e ragionevole. L'approvazione del subemendamento

che attiene necessariamente alle banche), che rimane con il credito insoddisfatto, perché spesso le somme, così ridotte a prezzo vile, servono a coprire i costi della procedura e incidono poco sul soddisfacimento del credito. Chi se ne avvantaggia, evidentemente, sono le manovre speculative, mediante le quali società o privati, in condizioni fisiologiche, si impossessano di beni immobili a un prezzo vile. Quando poi ci sono situazioni anche di tipo patologico (parlo di vicinanze a poteri criminali o di di disfunzioni, a voler essere generoso, di alcuni uffici giudiziari, delle sezioni fallimentari e delle esecuzioni immobiliari), questo ha un effetto ancor più dannoso e assolutamente ingiustificabile. Concludo dicendo che la tematica è di particolare importanza, al di là dei casi specifici, perché si inserisce nel contesto complessivo della gestione dei crediti non esigibili, con la notoria pressione degli istituti europei europei verso il sistema bancario italiano affinché questo si disfaccia dei cosiddetti NPL. Quello che sta avvenendo, anche mediante il sistema delle cartolarizzazioni, è il riversarsi sul mercato immobiliare italiano, tramite le aste fallimentari, di patrimoni per miliardi di euro, che stanno accedendo al mercato, con un crollo dei prezzi e con tutte le conseguenze negative del caso. Prendo atto del parere contrario; forse non c'è stata la possibilità e la capacità, da parte mia e di chi sostiene l'emendamento, di spiegare bene la giustezza della misura.

norme. Il voler intervenire con una norma così specifica nell'ambito delle procedure esecutive non risolve il problema che probabilmente si voleva andare a risolvere o c'era l'intenzione

La conversione del pignoramento (non so da quale testa sia stata partorita, sicuramente non da chi bazzica questo tipo di mondo) è uno degli istituti meno utilizzati in assoluto, perché un debitore non ha alcun interesse a mettere sul piatto tutti i costi della procedura (la casa, le spese, i creditori intervenuti), quando può farsi ricomprare l'appartamento da un prestanome ai tassi

anche alcuni aspetti legati alla procedura civile; non solo secondo me non era questa la sede, ma lo fa anche in modo assolutamente astratto. Mi

ci siamo associati qualche giorno fa, insieme con colleghi parlamentari, in occasione del secondo anniversario. Si tratta di una vicenda che si verificò in circostanze eccezionali. A quel tempo ero in Abruzzo, nel mio nel mio precedente lavoro. Ricordo le scosse e ricordo soprattutto l'eccezionalità delle precipitazioni nevose. Va anche detto però che a tali circostanze eccezionali e a questi eventi naturali, cui l'uomo non può, nella sua fragilità, opporsi, si aggiunsero forse episodi di gestione criticabili, censurabili, che non voglio evocare qui oggi e sui quali sono tuttora in corso delle indagini. Aggiungo anche un ricordo personale. A quell'epoca mai avrei immaginato di potermi esprimere in questa sede. Ricordo che pochi giorni prima ricevetti una telefonata dell'attuale ministro dell'interno Matteo Salvini, che mi chiese quale fosse la situazione e se fosse il caso di intervenire, di manifestare una presenza e una vicinanza. Poi lui intervenne ricordo che nel giorno immediatamente precedente alla tragedia Matteo Salvini e il collega Arrigoni erano lì, a Penne. Ricordo che ci furono

l'attuale Governo fa capire di avere un interesse reale e concreto per quelle vittime, di sentire il bisogno di riparare alla parte umana di quella tragedia, perché a quella naturale purtroppo non ci si può opporre. Sono fiducioso nel fatto che questo emendamento avrà un ampio accoglimento da parte di tutta l'Assemblea. *(Applausi

il coniuge rispetto al quale sia stata pronunziata sentenza «anche non definitiva» di scioglimento. Vi rendete conto dei problemi che si verranno a creare dal punto di vista delle successioni?

Certamente questo non risolve il loro dolore, ancora vivo. C'è un'inchiesta in corso a carico del prefetto di Pescara e di sei componenti della prefettura. Sicuramente, però, il Governo del cambiamento ha inteso intervenire, quantomeno per lenire il dolore

è stato espresso parere contrario a questo emendamento che chiede semplicemente di applicare la legge.

con tariffe che non scendono, visto che è scaduta la concessione autostradale, pur essendo ormai state pagate tutte le rate, diciamo così, per chi l'ha costruita. l'ha costruita. Addirittura non si vuole applicare la legge. Addirittura c'è un parere contrario all'ordine del giorno che impegna il Governo a farlo e la legge che lo stabilisce è il codice degli appalti. Volete cambiare il codice degli appalti? Tra l'altro è presente anche il Ministro competente, sia pure non nei nei banchi del Governo. Vogliamo proseguire? Si fanno i proclami contro le concessioni autostradali ma non bisogna essere né contro, né a favore, bisogna fare ciò che è giusto. Devono incassare il giusto e non troppo, e quando è scaduta la concessione - anzi, la legge dice due anni prima che scada la concessione - bisogna indire una gara, a meno che non si pensi che la competizione sia dannosa;

parere è contrario anche sull'ordine del giorno e nel frattempo centinaia di milioni al mese vengono incassati da privati quando le strutture sono di proprietà dello Stato.

tutte le autostrade - del nostro Paese sono di proprietà dello Stato, sia quelle gestite dall'ANAS, per intendersi quelle senza pedaggio, sia quelle con pedaggio. Il proprietario è lo Stato per cui sono un patrimonio dello Stato. Fino all'anno scorso, fino alla gestione precedente, era sempre stata pubblicata questa relazione, che è importantissima perché si parla di un giro di cinque o sei miliardi all'anno. Era sempre stata pubblicata al massimo a settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiva. Poi è arrivato il Governo del cambiamento, della trasparenza e questo elementare, doveroso momento di trasparenza non c'è. Ad oggi, siamo ormai a gennaio, siamo quattro mesi di ritardo rispetto alla peggiore data di pubblicazione precedente di questa normale relazione su come vengono spesi, come vengono impiegati, come vengono incassati questi sei miliardi all'anno che escono dalle tasche degli automobilisti italiani. automobilisti italiani. Gli si chiede di pubblicarlo almeno entro febbraio, cioè con soli sette mesi di ritardo rispetto agli esecrati Governi precedenti viene accolta come raccomandazione. Anticipo - così mi risparmio di intervenire dopo - che non accetto sia accolto come raccomandazione. È una cosa che è sempre stata fatta, si faceva per settembre, voi che siete il Governo del cambiamento, vi prendete sei mesi di più, ma si tratta semplicemente di mettere insieme dati raccolti da altri, non dovete assumere decisioni politiche,

Si tratta di due emendamenti molto importanti. Abbiamo condiviso in Commissione l'idea di eliminare tutti gli emendamenti che incidessero direttamente sul codice degli appalti.

Abbiamo pensato che la riforma del codice degli appalti dovesse essere fatta con un provvedimento *ad hoc* studiato, riflettuto, analizzato e ponderato. La riteniamo una buona legge, una nostra legge,

abbiamo votato contro tutti gli emendamenti, anche sensati, che incidessero direttamente sul codice. Per lo stesso motivo, però, abbiamo tenuto in piedi due emendamenti, appunto il 5.69 e il 5.71, che correggono delle modifiche fatte nel corso della legge di bilancio al codice, due correzioni *spot* e assolutamente, dal nostro punto di vista, errate. Il primo emendamento, il 5.69, è relativo alla centrale di progettazione,

al di sotto della quale sia possibile affidare appalti di forniture, servizi e lavori senza gare. «Un aiuto ai funzionari disonesti.

intervenire sul tema delle concessioni autostradali, perché è sempre bene distinguere ciò che è diverso e l'Autostrada del Brennero sicuramente

territoriali hanno così deciso di pensarla, progettarla e gestirla al meglio ed è tra le più efficienti e meglio mantenute d'Italia. in corso una trattativa molto importante tra gli enti territoriali, che sono naturalmente le Regioni, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la provincia di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Modena e Reggio Emilia e il

alla gara, secondo la direttiva e secondo le norme pubbliche. Da questo punto di vista, l'emendamento in esame mira a chiedere maggior tempo, perché questa trattativa difficile, ma che sta per diventare molto costruttiva con il Governo, possa arrivare a conclusione.

relativa all'anno 2016, perché quella del 2017, ad oggi - nel 2019 - non è ancora stata pubblicata dal nuovo Governo, mentre prima ci si metteva cinque mesi in meno. Tuttavia, anche su quei dati, che sono sicuramente più bassi di quelli di oggi, risulta che ad oggi sono già stati incassati dai concessionari 600 milioni di euro, solo nei mesi del nuovo Governo del cambiamento - lasciamo stare quelli prima - che legittimamente sarebbero dovuti entrare nelle casse dello Stato,

si faccia perdere tempo e dunque denaro allo Stato. Dunque viene certificato che, ritardando le gare o un affidamento di tipo diverso - *in house*, come è stato auspicato dalla senatrice Conzatti si perdano soldi. Dunque qui state votando per far perdere soldi allo Stato. Dandoli in beneficenza? No, dandoli a persone che, a quanto pare, non sono proprio tra i più bisognosi del Paese. Si tratta infatti dei detentori delle concessioni dello Stato, proprietà dei cittadini italiani, che, per fortuna e a merito loro, hanno delle aziende importantissime, che investono e hanno tanti soldi, anche all'estero.

si prefigge l'obiettivo di eliminare il Sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti (Sistri) e, nell'attesa che venga ideato un sistema elettronico alternativo, di ripristinare la tracciabilità del rifiuto cartaceo sulle regole previste dalla normativa esistente prima del 2010, anno in cui il decreto legislativo 205 ha apportato numerose e rilevanti modifiche al testo unico ambientale relativamente agli articoli 188, 189, 190 e 193. Tuttavia, i predetti articoli sono stati oggetto anche di modifiche apportate successivamente al 2010 proprio nello spirito di semplificare la normativa ambientale. Alcune di queste disposizioni sono ancora vigenti, poiché non abrogate, e attuali. Rischiano tuttavia di divenire inefficaci, atteso il fatto che nella nuova tracciabilità del rifiuto occorrerebbe applicare il testo previgente alle modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010. Con la proposta in questione si vuole, dunque, dare piena efficacia ad alcune semplificazioni introdotte dopo il 2010 e che, pur non avendo nulla a che vedere con il Sistri, con l'attuale formulazione dell'articolo in esame rischierebbero di venire disattese. Si tratta pertanto di un contributo alla semplificazione; ci viene dal mondo che opera intorno a questo settore. Chiediamo pertanto un ripensamento sul parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante

tutte le procure ci dicono che proprio sul traffico dei rifiuti la mafia si sta allargando e la cronaca ci racconta di molti episodi di incendi di depositi legali di rifiuti ma soprattutto di depositi illegali (capannoni o altro).

Gruppo PD)*. Presidente, questo emendamento, purtroppo, non è nelle condizioni di proporre un'alternativa al Sistri applicabile subito; quello che si può fare, però, è chiedere che a brevissimo - quindi, entro giugno il Governo provveda a introdurre un altro strumento di tracciabilità e di registrazione dei percorsi dei rifiuti per evitare che - ripeto -

prevedono ulteriori abrogazioni e alcune prescrizioni transitorie che intervengono anche sul cosiddetto codice dell'ambiente. Non è però previsto alcun intervento per recepire il parere S1062 del 29 luglio 2009 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con

di iscrivere nell'albo medesimo tutti quei professionisti che, in ragione della loro attività, effettuino operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi. Con l'emendamento in esame si raccoglie questo parere e si pone una regola al sistema.

Signor Presidente, stiamo parlando della gestione dei rifiuti speciali, che rappresenta un tema di estrema urgenza per il nostro Paese.

che è del tutto giustificato. È noto a tutti che gli impianti per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti speciali nel nostro Paese sono assolutamente carenti.

Dunque, è del tutto evidente la necessità che il trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non (pensate ad esempio a quelli sanitari), venga garantito, così come prevede la legge, all'interno di impianti abilitati e dunque certificati.

milioni di tonnellate all'anno - viene avviato allo smaltimento e, dunque, in alcuni casi in discariche autorizzate, oppure in impianti di termovalorizzazione. Che cosa si propone con l'emendamento in oggetto? Vista la carenza strutturale di impianti per la gestione di questi rifiuti nel nostro Paese, di lavorare in analogia con quanto previsto per gli impianti dei rifiuti urbani, ossia consentendo che vi sia la possibilità di operare a pieno carico termico fintantoché l'impiantistica nazionale non venga portata a regime e adeguatamente modificata e certificata. Questo emendamento però dice di più: l'impatto ambientale di questo pieno carico termico deve essere a zero. Esso quindi stabilisce una serie di normative, in particolare la certificazione EMAS e la certificazione OHSAS, relative sia alla certificazione ambientale che alla sicurezza del luogo di lavoro, affinché ciò possa avvenire.

il recupero energetico attraverso la termovalorizzazione di tutti i rifiuti, che siano rifiuti speciali o non speciali. Dunque chiediamo alla maggioranza un ripensamento. Sappiate - immaginiamo che tutti ne siano consapevoli - che la mancata assunzione di provvedimenti in questa direzione comporterà un impatto ambientale gravissimo

ritorniamo un'altra volta sull'annosa questione dell'*end of waste* che, lo ricordo, in italiano vuol dire «cessazione della qualifica di rifiuto», con cui ci si riferisce al processo di recupero eseguito su un rifiuto per farlo farlo tornare ad essere un prodotto. In questo momento - io lo sto ripetendo dal 6 marzo, insieme al Gruppo Forza Italia - le aziende di un comparto ambientale così importante rischiano la paralisi di uno stallo legislativo a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato che modifica le competenze rispetto all'ente che deve rilasciare le autorizzazioni (quindi anche in riferimento all'emanazione delle linee guida, perché ci sono delle direttive europee).

di non essere più l'unica voce che si leva. Al nostro emendamento, infatti, si era aggiunto quello della Lega, un emendamento del PD e persino un emendamento del MoVimento 5 Stelle, segno che la questione ormai è evidente e che il problema dei rifiuti che ci troveremo per strada, o in mano alla malavita organizzata o negli inceneritori tanto vituperati finalmente fosse stato compreso. Purtroppo, anche questa volta l'emendamento della Lega così come quello dei 5 Stelle sono stati prontamente ritirati, in nome del mantenimento di un'alleanza di Governo sempre più sottomessa ai compromessi in tema ambientale ed economico. Quindi ora è una pura scelta del Governo, anzi della parte gialla di questo Governo, che ha deciso di mettersi persino contro il proprio alleato, contro ogni evidenza. Non ne comprendiamo i criteri e quindi riteniamo che sia solo una precisa scelta e volontà politica quella di prendere tempo. Invece di tempo non ce n'è, perché le aziende rischiano la chiusura a causa del blocco degli impianti, i posti di lavoro diventano a rischio e la salute ambientale potrebbe essere compromessa per l'accumulo di rifiuti. Forza Italia rivendica il merito di aver sollevato la questione e di averla portata all'attenzione del Governo e del ministro Costa a più riprese, a partire dalle audizioni in Commissione. Continueremo a farlo in ogni provvedimento fino a che non sarà troppo tardi. Possiamo augurarci che questa insistenza serva quantomeno a sensibilizzare e a velocizzare l'azione del Governo. Non smetteremo di essere sentinelle. Non si può più perdere tempo, un tempo vitale per le aziende, per i lavoratori, per la salute pubblica. Un Paese povero di materie prime come il nostro non può permettersi di buttare in discarica o semplicemente bruciare i rifiuti e i prodotti a fine vita. *(Applausi dal Gruppo Signor Presidente, intervengo su questo emendamento, che poi è uguale al successivo, e ne approfitto anche per parlare di quelli che sono stati ritirati (ma l'intenzione di presentarli c'era comunque). Capisco la logica che sta dietro alla presentazione di questo emendamento, ma io vorrei pronunciare solo la seguente parola: CSS, ossia combustibile solido secondario. Nel momento in cui si scrive che una cosa cessa di avere la qualifica di rifiuto; nel momento in cui esiste un mercato per questa roba riqualificata ed è utilizzata per uno scopo specifico, allora il CSS, destinato alla co-combustione sia negli impianti di incenerimento che nei cementifici, ha un suo mercato e ha una sua classificazione merceologica. La buona intenzione va quindi temperata dall'idea di evitare che con una certa norma si possano fare delle cose che potrebbero non essere volute. Che la co-combustione in un in un cementificio sia una cosa che non presenta rischi per la salute purtroppo è smentito: i livelli di tollerabilità delle sostanze inquinanti nelle emissioni di un cementificio sono centinaia di volte superiori agli analoghi livelli assentiti per quanto riguarda gli inceneritori, i termovalorizzatori o come li vogliamo chiamare quando ci riferiamo agli impianti di distruzione termica della materia. Se lo scopo è quello di rendere utile un oggetto per un suo riutilizzo e possibilmente non un suo subciclaggio o una sua distruzione termica, allora questo tipo di proposta va fondamentalmente cambiato. Quindi, bene che la maggioranza l'abbia ritirato;

Presidente, è davvero inconcepibile, e per noi veramente incredibile, che la maggioranza non riesca a trovare un accordo su una questione così importante. Lo stesso ministro Costa aveva più volte ribadito l'urgenza di intervenire in questa materia e dunque di modificare le normative. Voglio ricordare che il Consiglio di Stato ha bloccato il rinnovo e le nuove autorizzazioni proprio autorizzazioni proprio a causa dell'assenza di un'adeguata normativa nazionale. È lo stesso Ministro che più volte ha invitato il Parlamento a trovare una soluzione. Non è possibile che l'incapacità da parte dei 5 Stelle e della Lega di trovare un accordo in tema ambientale stia non solo paralizzando questo Parlamento

sono mesi che fate delle baruffe chioggiotte pubbliche, spesso all'interno delle Commissioni o tra di voi, su un tema così importante. Non è più possibile attendere. I rifiuti speciali di cui parlavo prima non possono attendere, altrimenti entrano nel ciclo della mafia, dei roghi e degli incendi. L'*end of waste* non può più attendere per gli stessi motivi, e - aggiungiamo - perché c'è tutta un'economia circolare prevista dalla direttiva europea che attende di essere lanciata e che vuol dire conversione, posti di lavoro, qualità della vita, crescita della qualità dei nostri territori e quant'altro.

*a)* la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici; la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti; *d)* l'utilizzo «l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana». Questo prevede la normativa europea, che noi recepiamo con questo emendamento in un'armonica normativa nazionale. *(Applausi

Ripeto, l'alternativa è tornare in discarica (e in tutta Europa le discariche si chiudono, mentre in Italia si prorogano e si ampliano, in larghezza e in altezza)

è un bell'emendamento, che non ha oneri per lo Stato e dovrebbe essere condiviso anche da chi dei temi ambientali fa una bandiera. Esso nasce con la finalità di potenziare la vigilanza e le conseguenti azioni di bonifica dei siti di discarica abusiva sul territorio dello Stato, allargando l'azione del commissario straordinario nominato nel 2017 anche oltre gli ottanta siti assegnati perché colpiti da sanzione europea. Il risanamento dei territori avviene ora in maniera virtuosa secondo uno specifico schema organizzato e articolato, con una metodologia collaudata con un'apposita *task force* che l'Arma dei carabinieri ha affiancato al commissario per tali compiti. Questi criteri hanno creato una modalità di azione agile, efficace ed efficiente che ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di sanzione di 28 discariche abusive,

Pertanto, in considerazione delle argomentazioni che vi sto illustrando, questo *modus operandi* potrebbe essere applicato anche ad gli altri siti di discarica da risanare non colpiti da sanzioni dell'Unione europea (quindi operiamo in prevenzione non soltanto in emergenza)

Come ho ricordato prima, dal presente emendamento non derivano costi a carico dello Stato, perché le risorse da mettere a disposizione dell'Arma dei carabinieri non gravano sul bilancio dello Stato, ma verrebbero garantite attraverso un'autorizzazione a disporre di una percentuale non superiore allo

Signor Presidente, l'emendamento interviene in materia di fonti rinnovabili al fine di introdurre una disciplina che, in linea con i principi contenuti nella nuova direttiva sulla promozione dell'uso delle energie rinnovabili, assicuri certezza e perentorietà dei termini e degli *iter* autorizzativi per i relativi impianti, così da accelerare lo sviluppo degli investimenti necessari al raggiungimento dei *target* al 2030. Infatti, la presentazione della nuova strategia energia e clima da parte del Governo prevede che l'Italia si impegni a raggiungere una produzione da fonti rinnovabili su consumi finali pari a circa il 30 tale obiettivo determinerà un impegno economico-finanziario stimabile in oltre 60 miliardi di nuovi investimenti in impianti da fonti rinnovabili nel solo settore elettrico. Questo importante ciclo di nuovi investimenti negli impianti esistenti necessita quindi di tempi certi per i procedimenti autorizzativi. Si propone dunque di prevedere che l'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile debba essere rilasciata entro due anni dalla presentazione della relativa istanza e che debba includere anche la valutazione d'impatto ambientale. Inoltre, per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore a 150 chilowatt e per gli interventi di *repowering,* la durata del processo per il rilascio dell'autorizzazione non può eccedere un anno, salva l'estensione di un ulteriore anno in presenza di circostanze straordinarie.

il contratto di Governo assume un grande valore, perché quello che c'è scritto diventa vincolante, ha quasi valore di legge a sentire le ultime dichiarazioni di queste ore.

solo e ciascuno deve fare la propria presa. Questo emendamento, come l'articolo 8, è la presa dei 5 Stelle: in questa partita a carte la mano è dei 5 Stelle,

per l'Italia digitale viene messa direttamente sotto la Presidenza del Consiglio. I fondi vengono ridotti perché servono anche per fare una nuova società completamente pubblica. Questo è un decreto semplificazione e semplifichiamo aggiungendo una società in più, che ovviamente è a tutto favore della trasparenza. questa sia una questione da sottolineare perché in questo Paese stanno succedendo delle cose e tutte le cose che succedono e che riguardano la democrazia in questo Paese noi le andiamo a sottolineare: prendiamo l'evidenziatore e cerchiamo di far vedere, con un colore, che cosa sta succedendo. Per la prima volta abbiamo nel panorama politico una forza politica che dipende da una società di comunicazione una società di comunicazione che sta sviluppando una serie di attività in un momento nel quale la comunicazione, e la comunicazione digitale in particolare, assume un'importanza sempre maggiore, con tante implicazioni delle quali nessuno parla. In questi giorni, quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti a livello geopolitico mondiale: i Paesi stanno affrontando il tema della Huawei, ci sono lotte e battaglie, io direi quasi delle guerre sul tema della tecnologia, sul tema dell'accesso alle informazioni e di quanto a

però, è di mettere sotto la diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio un'agenzia. La Lega ovviamente non se ne interessa perché questa è la presa dei 5 Stelle. Noi, di fronte a questa opacità, a questa mancanza di dichiarazioni, di prospettiva e di chiarimenti sulla politica che vuole attuare questo Governo, diciamo:

il lavoro fatto negli anni precedenti, dai nostri Governi, ha dato dei risultati positivi, e ciò è implicitamente riconosciuto

Più volte è stato richiesto di superare il famoso vincolo della spesa legato diversi anni fa a più 1,4 per cento: tutte alchimie che non consentono alle Regioni che hanno le risorse di poter

vale per tutti: c'è chi governa oggi e chi governerà domani. Se la politica si vuole riappropriare della propria forza e del proprio

Un buon dirigente, di fronte a un indirizzo politico, deve indicare al politico la strada migliore per raggiungere l'obiettivo, e non la strada per dire: no, non si può fare; altrimenti che dirigente è?

poi - questo è un impegno che prendiamo come Parlamento - la risposta deve essere sì: superiamo questo vincolo che sta mettendo il Paese in grosse difficoltà e che vale per tutte le Regioni, da Nord a Sud. *(Applausi dai

ci sono, oppure non ci sono. Ci sono delle procedure e delle norme che, presidente Romeo, vanno necessariamente rispettate. Se qualcosa non funziona, non si usa l'Assemblea parlamentare per fare delle minacce ai dirigenti dello Stato che fanno il loro lavoro. Io prego il presidente Romeo di ascoltare bene quello che ha detto, annunciando certe future decisioni e certe future attenzioni da parte della maggioranza. Quindi, la mia richiesta a questo punto, rispetto all'istanza molto chiara del presidente Romeo, è che venga il ministro Tria a riferire su cosa sta accadendo, perché le dichiarazioni del presidente Romeo sono assolutamente gravi e molto pericolose per il funzionamento di questo Parlamento. Allora io chiedo che venga il ministro Tria e chiedo che il Presidente metta ai voti tale richiesta, perché a questo punto le dichiarazioni e le parole sono pietre e hanno un loro peso specifico. Chi ha parlato non è un parlamentare qualsiasi, è il Presidente del Gruppo di maggioranza determinante su questi passaggi parlamentari. Quindi, non possiamo semplicemente ascoltare e fare finta di niente; vorremmo anche sapere cosa pensa il presidente Patuanelli di questa vicenda. Quindi, la richiesta del Partito Democratico,

che vi sono altri due sbarramenti (il fondo e il rispetto del fondo), allora non serve fare delle minacce. Il Governo ci proponga un atto. Senatore

pasticciato e confuso in relazione alle competenze, perché la competenza organizzativa del personale è esclusiva delle Regioni.

Adesso facciamo il nostro mestiere: presentiamo un subemendamento e superiamo il vincolo dell'1,4

cancelliamo il vincolo dell'1,4 per cento, impegnando il Governo a presentare al più presto

è di tutte le Regioni, perché quelle in maggiore difficoltà e che hanno bloccato il personale in quei termini sono all'emergenza, prima di tutto al Sud. E questo è un problema che ci riguarda pesantemente.

accolgo veramente con entusiasmo l'intervento del capogruppo Romeo, perché per due settimane io e il collega Vitali ci siamo agitati in Commissione esattamente per la stessa, identica cosa. Ogni volta

di poter gestire quel tipo di provvedimento che si sarebbe approvato - e si trattava di tutta una serie di emendamenti che avrebbero influito sulla buona organizzazione delle Regioni e degli enti locali attraverso responsabilità dirette dei dirigenti.

evidenzia esclusivamente una confusione generale all'interno della maggioranza: la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra; o meglio, le due mani di sinistra non sanno cosa fanno l'una rispetto all'altra, perché questa è la condizione in cui oggi versa la maggioranza. versa la maggioranza. La questione è molto importante, perché bisogna capire fino in fondo se l'esercizio di maggioranza deve essere espletato fino alla fine. Nella mia esperienza da amministratore ho fatto approvare dalla mia giunta e dal mio consiglio comunale una sequenza enorme di provvedimenti col parere contrario degli uffici, perché avevo ben chiaro che l'obiettivo politico dell'interesse della mia comunità sarebbe stato esattamente il contrario di quello che gli uffici in quel momento mi stavano dicendo. Quindi, se la maggioranza ha gli attributi per essere dichiarata tale, l'emendamento in questione, anziché votarlo come ordine del giorno, che vuol dire aria fresca, si approva così com'è e ci si assume la responsabilità fino in fondo del rapporto con gli uffici. Se un consiglio comunale dipende da vari altri organismi superiori, il Senato e il Parlamento sono sovrani rispetto a tutti gli organi dello Stato, e di conseguenza

punto di vista di qualsiasi dirigente, il quale si dovrà per forza adeguare. Siate quindi conseguenti e non ipocriti.

perché sono convinto che negli ultimi anni è andato avanti un processo degenerativo che è continuato e si è dilatato, all'interno del quale la politica è stata lateralizzata. Il primato della politica si è perso, perché altri poteri dello Stato hanno svolto attività sostitutiva o di supplenza del tutto impropria. Qui mi fermo, senatore Romeo. Un conto è questa affermazione; un conto è il ruolo

di andare avanti e il consiglio comunale ha votato. Lei non si è deresponsabilizzato, ma si è assunto la responsabilità politica

il Ministro dell'economia - viene, ci mette la faccia, si assume la responsabilità e non scarica

per mandare messaggi obliqui alla Ragioneria generale dello Stato. Questo non fa onore a lei e neanche al Parlamento. Non è il ruolo del Parlamento. Diverso è il discorso, teorico, di principio, di cui - lo condivido - dovremmo parlare. Penso che avremo occasione per farlo e allora vorrò vedere se la maggioranza applaudirà, come ha fatto oggi quando si è parlato di primazia e di primato della politica.

il ragionamento che il presidente Casini ha iniziato a sviluppare in Assemblea ha sicuramente dignità di proseguire, brevemente adesso, ma probabilmente in modo più

ha esercitato questo suo ruolo più come una supremazia che come un primato, a prescindere dal mandato elettorale ricevuto. Credo che i conflitti che noi oggi valutiamo tra la politica e

inadeguata ad assumere certe decisioni e dopo una stagione, quella di Tangentopoli, che ha portato alla legge Bassanini, che ha dato molto potere a quella classe dirigente che oggi

ai cittadini che hanno fatto una scelta votando delle forze politiche. Mi ricollego a quanto diceva il presidente Romeo: in fondo il tema è questo. Noi abbiamo preso degli impegni con i cittadini e vogliamo portarli avanti. Vale per questo emendamento, ma vale, in generale, per le elezioni politiche che questa questa maggioranza e questo Governo stanno cercando di portare avanti. A prescindere dal parere di un tecnico, quindi, se c'è la volontà politica di portare un'azione politica in una direzione, il Parlamento deve essere in condizioni di farlo. Credo che su questo occorra una riflessione comune, e la faremo in altri momenti perché necessaria. Per ora, però, mi allineo alle parole del presidente Romeo quando dice che questo emendamento diventa un ordine del giorno, ma non è un ordine del giorno scritto - come si usa dire -

d'importanza assoluta, perché le democrazie si reggono anche sul principio sacrosanto del primato della politica e io penso che su questo tema

fatto non soltanto nel nostro Paese, ma in tutte le democrazie occidentali. Vorrei però fare un'osservazione sulle dichiarazioni del senatore Romeo, che mi sembra riguardi anche l'intervento del senatore Patuanelli, perché anche la politica, pur esercitando il suo primato, deve conoscere i limiti della sua azione. Il senatore Romeo ha fatto riferimento agli organismi tecnici che sovrintendono al bilancio dello Stato. Vorrei solo ricordare, perché il Parlamento ne abbia memoria, che c'è stata una fase della vita del nostro Paese in cui la politica ha esercitato il proprio primato e lo ha fatto in contrasto con le indicazioni le indicazioni tecniche degli organi dello Stato e in tale fase il Paese ha fatto 2.300 miliardi di euro di debito pubblico.

La politica ha quindi il dovere di esercitare il suo primato, ma deve sapere che lo deve fare all'interno di quella regola, che indica indica che per ogni euro che destiniamo a qualche obiettivo che riteniamo meritevole deve esserci un euro che entra, perché il bilancio dello Stato ha bisogno di un equilibrio non diverso dal bilancio delle nostre famiglie

e soprattutto dell'autorevolezza e del prestigio che negli ultimi anni abbiamo perso. Visto che i presentatori sono tutti componenti delle Commissioni riunite, senza che questo costituisca un precedente, ha facoltà di parlare anche il senatore Bagnai,

il dibattito che si è aperto è molto interessante e concordo con il collega Zanda sul fatto che meriterebbe tempi più distesi che non possono essere questi. Se mi permettete, però, di fare un momento il professorino, vorrei aggiungere due precisazioni che credo ci aiutino a focalizzare il problema. Intanto, mi è sembrato di sentire assimilare la Ragioneria generale dello Stato ad un'autorità indipendente. Non credo che sia esattamente così. Non tutto quello che è tecnico è indipendente, anche perché la tecnica ha perso

secondo me, dovrebbe essere un pochino riconsiderata. Gli individui nascono, muoiono e lasciano un'eredità. Lo Stato - diciamo così - non muore ed è il luogo dove si esplica la solidarietà anche intergenerazionale: l'idea che per un euro che entra debba uscire un euro o che per un euro che esce debba entrare un euro è molto statica, molto povera. Sono sicuro che il collega Zanda abbia un bagaglio culturale che gli consente di avere una visione un pochino più ampia del processo macroeconomico. Basti osservare una cosa,

Mi pare che nessuno abbia contestato interventi anche importanti. BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Vorrei far notare che l'Italia ha un passato di avanzi primari importanti. Il motivo per il quale il debito è esploso è un pochino più complesso del non aver esercitato la diligenza del buon padre di famiglia Grazie

Commissioni riunite per capire che cosa portare a casa per il comparto sanità e credo che questa notizia davvero sia ferale. Ritengo si debba intervenire il più presto possibile attraverso un emendamento, come detto dai colleghi, per sanare una situazione che ormai è insanabile, anche perché su questo provvedimento, il decreto semplificazioni, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Devo ringraziare il Presidente del Senato che ha fatto ritirare emendamenti che andavano a toccare la vita delle persone come anche la libertà individuale: ricordo a tutti che abbiamo rischiato di complicare ulteriormente le dichiarazioni anticipate di trattamento, che avevamo portato a termine nella precedente legislatura, una mano, nella notte, voleva approvato un emendamento per complicarle ulteriormente. Grazie a Dio l'emendamento è stato ritirato, ma era un altro rischio per la libertà

semplificando, a mio parere, ed ecco perché questo emendamento. Fino al 2021, è possibile dare incarichi a chi sta facendo formazione, ancorché non abbia terminato la sua formazione completa, dandogli la possibilità di accedere ad un bando di concorso per medici in formazione. Il fine di questo emendamento, di avere un decreto che stabilisca un'omogeneità di formazione in tutto il Paese, ovviamente in accordo con le Regioni, perché la formazione per i medici di medicina generale è a carico delle Regioni. Dico questo perché noi abbiamo bisogno che tutti i medici di medicina generale, come in tutte le specializzazioni, abbiano un *unicum*, un *core business*, un *curriculum*, in modo tale che tutti abbiano lo stesso tipo di formazione. Questa è una cosa importante che non è stata considerata. È stato approvato un mio ordine del giorno in Commissione sanità, perché tutti eravamo d'accordo sul punto, bellamente, è stato dato parere contrario. Anche quello della medicina di emergenza-urgenza è un tema importantissimo, che tocca tutti noi in quest'Aula: senza medici in pronto soccorso noi non possiamo essere sicuri in nessun luogo, neanche qui dentro. È un allarme che arriverà sicuramente da questo

che ha annunciato poc'anzi in Aula. Credo che il tema sollevato sia rilevante e ricordo ai Capigruppo di maggioranza - ad entrambi i Capigruppo di maggioranza - e al Governo tutto che la nomina del Ragioniere capo dello Stato è una nomina di responsabilità collettiva: su proposta del Ministro competente, il Ragioniere capo viene nominato dal Consiglio dei ministri, che vota e, nel momento in cui ciò avviene, il Governo nella sua completezza e nella sua collegialità e, di conseguenza, la maggioranza parlamentare che lo sostiene, si assumono delle responsabilità e si fanno carico delle responsabilità che questa persona - che tra l'altro considero autorevole - andrà a svolgere. Allora mi domando quale sia il significato dell'attacco che ha fatto il presidente Romeo rispetto alla Ragioneria generale dello Stato: è un atto di sfiducia da parte della maggioranza parlamentare nei confronti di chi dirige la Ragioneria generale dello Stato? è una domanda e aspetto risposta. È un atto di sfiducia nei confronti del Ministro, che ha proposto questa nomina al Consiglio dei ministri? un atto nei confronti del Governo nella sua globalità? Ce lo deve spiegare, presidente Romeo, perché noi, rappresentanti del popolo in quest'Aula, abbiamo il diritto di capire cosa ci ha detto, perché i messaggi obliqui - mi permetta - non sono consoni a quest'Aula. Qui abbiamo diritto alla trasparenza e alla comprensione. *(Applausi comprenderanno tutti i cittadini cosa sta dicendo. Si sta riferendo a manine del passato, che qualcuno ha trovato in alcuni provvedimenti, oppure ad altri atteggiamenti? Eppure, per alcuni provvedimenti importanti, alcuni dei quali non condivido affatto, nei contenuti e nelle conseguenze

Signor Presidente, quello in esame è un ordine del giorno scritto male, dovuto non so se ad un momento di isteria o ad una presa di posizione politica rilevante. È inaccettabile che ci si comporti in questo modo ed è inaccettabile che il Senato venga trattato così. MALLEGNI *(FI-BP)*. Leggilo! sanno cosa hanno scritto in questo ordine del giorno. Dopodiché, siccome nel merito siamo d'accordo sull'emendamento originario, nel merito eravamo d'accordo in Commissione e lo siamo anche in questa sede, chiediamo al Governo - noi sì di rispettare la volontà del Parlamento: di trovare i fondi e di andarli a prendere, magari da quelle misure pericolose che avete voluto approvare e finanziarie e che mettono a rischio il nostro Paese per il futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Diamo delle risposte concrete e serie alle esigenze dei cittadini italiani! Andiamo a lavorare sulla loro salute e non usiamo il Parlamento per dare messaggi obliqui e per fare delle minacce, perché non è questa la sede. Le minacce, presidente Romeo, le deve fare altrove, le deve fare nelle riunioni di maggioranza, non le deve fare utilizzando il Senato

ci chiarisca il significato delle parole del presidente Romeo e la loro portata, se è o non è un atto di sfiducia della maggioranza parlamentare nei confronti del Ragioniere capo e nei confronti del Ministro, la cui presenza reputo ancora ora necessaria in quest'Aula.

legge, che vanno tutelate e garantite, perché sono un elemento di equilibrio e la democrazia è sempre un tema di equilibri. Detto questo, chiedo ai relatori se vogliamo davvero affrontare la questione - di cambiare l'ordine del giorno in esame. Questo ordine del giorno non risolve il problema, cambiamolo, scriviamo: «si impegna il Governo, in un prossimo

il problema non è relativo alla copertura: per quel che riguarda il personale, non c'è un problema di tale tenore, perché il fondo sanitario nazionale non ha il vincolo sul personale;

timbro, sotto questo profilo, se si pongono le questioni in modo corretto, senza scaricare le responsabilità sugli altri. Chiedo quindi, veramente, ai relatori

riteniamo doveroso e opportuno generare le condizioni affinché si perfezionino i contenuti dell'ordine del giorno che è stato presentato dai relatori.

ognuno per quanto riguarda le proprie competenze, è necessario infatti traguardare un cambio di paradigma che sia autenticamente vocato ad una responsabilizzazione, ma anche ad una semplificazione dei processi sia di riqualificazione della spesa sanitaria,

le condizioni perché tutti i sistemi sanitari regionali possano finalmente superare i lacci e i lacciuoli di un vincolo che affonda le proprie radici ad oltre quindici anni

da dieci anni non avevano il contratto di lavoro rinnovato per vari blocchi e varie difficoltà. Ovviamente, questo sta causando l'impoverimento di medici nel Sistema sanitario nazionale, che che cercano migliori occasioni nel privato e spesso emigrano all'estero, impoverendo il Sistema sanitario nazionale anche in senso qualitativo.

porta, nella area contrattuale dei medici e dei dirigenti propriamente sanitari, altri dirigenti, altre figure, quali

dei turni, non hanno il vantaggio dell'esclusività di rapporto. Questo, da un lato, rischia di incrementare addirittura le spese, perché farebbe accedere a determinati benefici categorie che non avrebbero motivo di averne; dall'altro lato, però, inserisce queste figure - 5.000 fra avvocati, ingegneri e personale tecnico competente e fondamentale per il buon funzionamento del Servizio sanitario nazionale - in una platea di 150.000 dirigenti, dirigenti, impedendo a queste persone di avere rappresentanti che, a livello nazionale, vadano a contrattare il loro contratto di lavoro, entrando nel contratto di dirigenti con altre caratteristiche. subemendamento - che, purtroppo, è stato respinto - era volto a richiedere un'area contrattuale specificamente dedicata a questi dirigenti, fondamentali anch'essi per il buon funzionamento del servizio sanitario pubblico.

2011, e dei presidi incaricati al nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di dirigente scolastico, per sanare il contenzioso in corso, giunto già dinanzi alla Corte costituzionale, sulla legittimità della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle successive assunzioni disposte. Non vi sono oneri finanziari. Si tratta di sanare una disparità di trattamento tra due categorie messe a concorso. Vi è un contenzioso lungo, che si protrae da anni e sta per arrivare dinanzi alla Corte costituzionale. Durante le audizioni svolte nelle Commissioni riunite abbiamo ascoltato tutti i rappresentanti delle categorie interessate e da tutti è pervenuta, in maniera unanime, questa richiesta. Quindi, non si capisce per quale motivo non si voglia accogliere, quanto meno per un principio

da 87 a 90, ha previsto la possibilità, per alcune categorie di concorrenti delle procedure concorsuali del 2004, del 2006 e del 2010, di partecipare a una procedura riservata (decreto direttoriale n. 499 del 2015), operando una grave disparità di trattamento verso i ricorrenti del

in vigore della legge n. 107 del 2015. Ciò non ha consentito loro la partecipazione alla procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata. Ricordo a quest'Aula che che vi sono 2.000 sedi vacanti per dirigenti scolastici e che ogni anno si ricorre alle reggenze provvisorie, con grave nocumento per gli stessi dirigenti scolastici, costretti a dividersi

La norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del dirigente scolastico, le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell'istruzione e della ricerca. Dall'applicazione si prevedono risparmi da stornare nel Fondo di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° marzo 2002, a seguito dell'approvazione del contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016. Per il triennio 2015-2018 erano stati stanziati 7 milioni di euro all'anno. Chiediamo un ripensamento sul parere dato a questo emendamento con una disposizione favorevole al suo accoglimento.

la cosiddetta terza missione. Tutti sappiamo che le università hanno due missioni molto precise: la ricerca e la docenza. Però da molto tempo l'Anvur considera particolarmente importante il dialogo tra le università, la società, la società, il mondo del lavoro, le imprese; lo considera e lo valuta in termini di brevetti, di consulenze, di un'azione discendente nel senso di professori universitari che fanno formazione sul campo nelle aziende; e viceversa, professionisti che entrano nelle università, e a loro volta portano l'esperienza della società civile all'interno dell'università. Questa complessa rete di attività che va sotto il nome di terza missione è esattamente quella rappresentata in questo emendamento che di fatto è già una prassi perché l'Anvur, quando valuta le università, le valuta anche sotto questo profilo. Aver proposto questo emendamento, che mi piace anche sottoscrivere, significa aver posto in chiave normativa quello che, di fatto, sta diventando prassi. Io credo che bocciare questo emendamento significa in realtà mandare un messaggio del tutto negativo non solo alle università, ma anche a quell'organismo sovracostituito, che è l'Anvur, previsto esattamente come strumento di valutazione dell'università e della ricerca. Mi risulta praticamente ridicolo che un emendamento a costo zero - perché non esiste nessun costo su questo, ma semplicemente una formalizzazione di processi e procedure - sia stato bocciato.

Da molto tempo, da quando non c'è più un Ministro dell'università e della ricerca, l'università è veramente la Cenerentola. Lo dimostra il fatto che sono stati bocciati tutti gli emendamenti che vanno in direzione del miglioramento della vita universitaria, ivi compreso - e mi permetta di dirlo - un emendamento altrettanto a costo zero che, essendo stato bocciato, corre il rischio di mortificare profondamente e di complicare la vita delle facoltà di medicina. Infatti, essendo stato approvato, finalmente, dopo tanti anni, l'esame abilitante di medicina, l'emendamento chiedeva che non entrasse in vigore a luglio, ma semplicemente nel 2020.

ci capiamo), è funzionale al messaggio che il Presidente del Senato ci ha dato nella giornata di ieri. Ci sono tantissimi interventi urgenti, tante questioni che riguardano la semplificazione, che abbiamo dovuto mettere da parte e che finiranno in un disegno di legge

non deve essere un *omnibus*. Sia chiaro che questo è il motivo, non ci sono altre questioni. Nel merito saremmo anche d'accordo, come abbiamo fatto per tanti altri emendamenti. Lo ritiriamo, ma è importante capire che il tema sarà inserito, poi, in un disegno di legge.

l'emendamento 10.0.11 (testo 3). In particolare, il punto 3 è molto interessante, perché per la prima volta si pone l'accento sul fatto che in Italia non ci sono abbastanza borse di studio per dottorati di ricerca.

Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 10.0.1000/2 che cerca di attenuare o di correggere alcune conseguenze molto negative dell'emendamento del Governo, che rappresenta peraltro un classico esempio di cattivo legiferare,

perché alla fine di dicembre, nel corso delle contestazioni che a giorni alterni vedevano contrapposti tassisti o NCC, il Governo ha deciso di espungere dal testo della legge di bilancio una norma che riguardava gli NCC, promettendo di varare un provvedimento *ad hoc* da inviare al Parlamento in modo che ci fosse tutto il tempo di discuterlo e di approfondirlo. Così è stato, infatti il Governo ha approvato un decreto-legge, lo ha inviato alla Camera, che ha iniziato a svolgere le audizioni, ha sentito le parti improvvisamente, inopinatamente, quel provvedimento è stato riversato integralmente come emendamento all'interno di questo decreto-legge semplificazione che, come stiamo vedendo, di semplificazione ha sempre meno.

annullate ogni principio di libera concorrenza, di mercato, colpite un settore che non è fatto solo da Uber o dalle grandi società, ma da padroncini, da lavoratori autonomi da gente disperata che ha speso soldi per acquistare

mettendo a rischio il futuro dei loro figli. Ieri erano stesi qui davanti al Senato - devo dire anche caricati eccessivamente dalle Forze dell'ordine, che hanno sempre il mio grande rispetto, ma ieri a mio parere hanno esagerato - solo per dirci che questo provvedimento li distrugge, li mette nelle condizioni di non lavorare più. Questa è una responsabilità fortissima che il Governo si sta assumendo, per cui il Partito Democratico voterà assolutamente contro. Per questo mi piacerebbe vi fosse un ripensamento da parte delle forze di maggioranza e per adesso lascio agli atti il mio intervento e la volontà del Partito Democratico di fare fino in fondo la propria parte

Forse abbiamo la responsabilità - parlo della politica - di aver messo contro due categorie di lavoratori che sono e debbono essere necessariamente rispettate entrambe. a nostro parere, perché l'Italia è un grande Paese e ha necessariamente sfaccettature diverse perché il centro di Roma è sicuramente diverso dal centro del Comune di Pietrasanta, mi sembra evidente. A Roma ci sono migliaia di licenze taxi e qualche centinaio di licenze NCC. Nel mio Comune sono state rilasciate diverse decine di licenze NCC e qualche licenza taxi taxi perché il servizio è diverso, la funzionalità è diversa e non si fanno assolutamente la guerra gli uni con gli altri. L'Italia non è solo Roma.

perché non rendiamo un servizio alla gente che lavora. Entrambe le categorie hanno il diritto di lavorare e di guadagnare. Noi ci siamo permessi di presentare un emendamento

evidenziando che esistono Città metropolitane e che esistono paesi e città in cui la problematica del rapporto taxi - NCC non c'è. Noi dobbiamo sapere cosa serve al turista, cosa serve al cittadino, cosa serve al commercio, non se abbiamo amici che hanno la licenza NCC o se hanno il taxi, a seconda dei voti che danno all'uno o all'altro. Ma la facciamo finita? Ma che servizio rendiamo a questo Paese? Dobbiamo sapere che abbiamo 320.000 alberghi, 30.000 imprese balneari, centinaia di migliaia di negozi che hanno bisogno che le persone vengano accompagnate

se la maggioranza del Parlamento volesse apporre la propria firma saremmo ben lieti di accoglierla perché sarebbe veramente un bel gesto nei confronti delle imprese che lavorano. In questo emendamento identifichiamo le problematiche delle Città metropolitane e garantiamo i taxi, diciamo che c'è un'altra Italia e garantiamo tutti.

Democratico sulla manifestazione di ieri dinanzi al Senato. Pur comprendendo lo stato d'animo di chi ha manifestato, tutto il Gruppo Forza Italia vuole ribadire che noi siamo sempre dalla parte delle Forze dell'ordine, che ieri hanno avuto l'intelligenza e la lungimiranza di non portare feriti gravi, nonostante siano state lanciate delle bombe carta. Ringraziamo le Forze dell'ordine per la saggezza e la lungimiranza con cui hanno gestito ieri l'ordine pubblico davanti al Senato.

Ritengo sia in atto una guerra da parte del ministro Toninelli nei confronti del territorio, che va da Modena al Brennero, perché la società in questione ha fatto "i compiti a casa",

La smetta quindi Toninelli di fare il bambino, provveda al rinnovo della concessione, perché quel territorio ha bisogno di quelle ingenti risorse. *(Applausi

spendono non 100.000 euro, non 30.000 euro, ma 25.000 euro al chilometro. Quindi è gestita bene, ha un programma di investimenti trentennale

e che vuole mantenere le promesse fatte al territorio, dal Brennero a Modena, di investire e di gestire bene l'impianto autostradale.

di un emendamento molto importante, che forse avrebbe meritato un voto favorevole, dato che ne abbiamo discusso moltissimo in Commissione e l'apprezzamento di un ordine del giorno

(e mi riferisco appunto alla concessione sull'autostrada A22). Con la trasformazione in ordine del giorno si chiede il recepimento della Direttiva 2014/23/UE, con particolare riferimento

riflettere tutti ancora una volta: come vedete, questo è esattamente il provvedimento che sta alla Camera. Mi meraviglio molto che sia stato reso ammissibile; mi meraviglio molto - e lo sottolineo due volte

risolvere e governare i problemi che si sono creati; è solo un modo per continuare a contrapporre due categorie. Quando al milleproroghe - il relatore Collina se lo ricorderà perfettamente - fu presentato un emendamento,

da almeno dieci anni poiché non si vogliono affrontare. Sarebbe stato giusto proseguire l'*iter* iniziato alla Camera, perché questo avrebbe comportato la possibilità di costruire un dialogo e di riuscire a trovare

tassisti. Per questo bisognava intervenire per trovare un equilibrio e non forzare come si sta facendo. Per tutti questi motivi, voteremo contro come senatori di LeU e Gruppo Misto.

che non abbiamo fatto niente in questi mesi. Ha fatto bene la senatrice De Petris a ricordare che negli ultimi dieci anni non si è fatto niente è approdata qui, sul tavolo, in tutta la sua violenza. Io l'ho portata all'attenzione delle Commissioni riunite e ne ho parlato molto chiaramente. il piacere di poter ricevere, per la prima volta, le categorie sia dei taxisti che degli NCC. Sono consapevole nel dettaglio

alleggerire una posizione che era controversa da anni. Oggi gli NCC non devono più rientrare alla base; possono prendere le chiamate telefonicamente. Fare un intervento un po' più complesso e completo significa mettere mano a un compendio normativo e sarà nostra premura farlo.

Quale esempio darebbe la politica oggi a questi giovani che, con preparazione, con ardore, con i valori, vogliono vestire la divisa della Polizia di Stato? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Non è giusto e non è corretto; sarebbe un cattivo esempio. Mi appello pertanto a quella forza politica affinché possa ritirare questo emendamento e quindi i giovani oggi possano aspirare a un valoroso posto di lavoro.

nella discussione generale da più parti è venuta un'istanza pressante, nei confronti della maggioranza e del Governo, di rivedere questa posizione. Un'istanza pressante che deriva dalla mobilitazione di migliaia di ragazzi che con questo emendamento verrebbero eliminati dal raggiungimento di un obiettivo del quale hanno fatto il punto di riferimento della loro vita. Signor Presidente, non è tanto o solo importante il fatto di togliere la speranza e la possibilità a questi ragazzi che hanno fatto un concorso,

il problema è di varare una norma con effetto retroattivo che è assolutamente incostituzionale e che urta contro tutti i principi di legittimità *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*, indipendentemente se si tratta del concorso di Polizia o di qualunque altro concorso. concorso. Uno Stato serio non può chiedere il rispetto di determinati requisiti e, dopo aver espletato il concorso, eliminare una parte di questi requisiti. Si tratta allora di giustizia per questi ragazzi, ma si tratta di buon senso da parte della maggioranza e del Governo. Noi ci auguriamo che ci sia un ripensamento, ma in ogni caso chiediamo che sul punto qualcuno ci dia una risposta. Ci dica il perché di questo emendamento. O si ha il coraggio e il senso di responsabilità di ritirarlo, oppure si abbia il coraggio di assumersi le proprie responsabilità in Parlamento e dire quali sono le ragioni, anche recondite, che portano alla presentazione e al voto di questo emendamento.

Signor Presidente, colleghi, questo emendamento ieri era dentro l'elenco di quelli considerati improponibili. Solo dopo qualche minuto la Presidente, la cui espressione è insindacabile, ha detto che la presenza dell'emendamento 11.17 (testo 4) all'interno di questo elenco era da considerarsi un errore. Presidente, sono abbastanza convinto del fatto che è un emendamento che darà vita alla seguente situazione. Colleghi, scusate se torno sul tema già ieri posto in discussione generale, ma sono convinto che la vostra indifferenza non sarà la risposta a questa votazione. Nella medesima graduatoria di un concorso del 2017

un'età, un titolo di studio e una prova superata. Voglio sapere come facciamo ad approvare un emendamento che cambia oggi questi requisiti. Non lo possiamo fare.

«Non ci possiamo fare nulla». Voi sapete che stiamo assumendo un atto illegittimo. È evidente che non è questione di diritto; non si possono cambiare i requisiti in corsa. Aggiungo - se qualcuno della maggioranza avesse la disponibilità a interloquire - che non vale obiettare che i requisiti sono stati cambiati nella scorsa legislatura, a luglio 2018. Infatti, a novembre 2018, ossia dopo la modifica della normativa, da questa stessa graduatoria sono stati chiamati i ragazzi

dopo la modifica cui si fa riferimento, ancora si utilizzano i vecchi criteri. Oggi, per la prima volta, introduciamo il criterio dell'attingere in maniera selettiva alla medesima graduatoria. Credo non si possa fare e chiedo chiedo ai relatori del provvedimento in esame di considerare l'illegittimità di ciò che stiamo facendo e di non calpestare non solo i diritti, ma anche i sogni di questi ragazzi. Prego senatore, il voto favorevole sull'emendamento 11.17 (testo 4), che è complesso e articolato e comprende varie semplificazioni da apportare nell'ambito di interesse dell'attività del Ministero dell'interno. Concentro questa mia breve dichiarazione sull'inserimento del comma 2-*bis*, quello su cui, come abbiamo appena visto, si è maggiormente concentrata l'attenzione politica e mediatica. Vi è innanzitutto la necessità di provvedere a reintegrare, nel minor tempo possibile, un consistente numero di agenti di Polizia di Stato per far fronte al mancato *turnover*, conseguenza del vostro blocco delle assunzioni *(Applausi

di contrasto all'immigrazione clandestina e al terrorismo internazionale. Non agire tempestivamente e con coraggio, avrebbe voluto dire accodarsi alle azioni del Governo precedente, che ha via, via smantellato l'organico *(Commenti dal Gruppo PD)*, con la conseguenza di portare alla soppressione dei piccoli commissariati e alla progressiva chiusura di reparti, quali quelli della Polizia ferroviaria, della Polizia postale e della Polizia stradale.

Anziché procedere alla lunga e costosa indizione di un nuovo concorso, si prevede di utilizzare gli esiti parziali di quello recentemente svolto nel 2017, attingendo dall'elenco dei candidati che, seppur non ottenendo l'idoneità finale, hanno superato positivamente la prova scritta, adottando quindi criteri decisamente meritocratici. Tale nuova procedura semplificata e sostitutiva di un nuovo concorso e dei relativi costi (e non è la prosecuzione di quel concorso) trova però a scontrarsi, come detto, con quanto previsto dal decreto di riordino delle carriere, approvato nella scorsa legislatura dalla precedente maggioranza. I requisiti più rigorosi relativi al titolo di studio e all'età massima non vengono, quindi, stabiliti dalla nostra azione emendativa, ma sono l'eredità di scelte precedenti. Non adottare questi requisiti avrebbe significato far venir meno il principio di equiordinazione con le altre Forze, che nel corso di questo stesso anno avvieranno concorsi con i nuovi requisiti. La scelta di tale percorso avrebbe quindi reso illegittimo e vano lo scorrimento totale della graduatoria, a discapito di tutte le categorie di partecipanti e della sicurezza pubblica. Come Gruppo Lega abbiamo quindi presentato e sosteniamo convintamente questo emendamento, perché siamo certi di non ledere alcun diritto acquisito.

procedere celermente a garantire più sicurezza ai territori e ai cittadini Signor Presidente, intervengo per dire che il Gruppo Forza Italia non solo è a favore delle assunzioni dei 1.800 poliziotti, ma anzi ritiene che dovremmo fare molto di più perché gli organici sono assolutamente sottodimensionati *(Applausi un Governo della scorsa legislatura con il ministro Madia, colleghi del PD, dispose anche una riduzione definitiva e stabile delle piante organiche delle forze di polizia, facendo un grave errore, perché le adeguò alla ristrettezza di personale, invece avrebbe dovuto

dal Gruppo FI-BP)*: meglio creare posti di lavoro nella sicurezza che finti redditi di cittadinanza o altre cose da cui siamo sommersi

che queste persone vengano prese in tempi rapidi proprio per metterle a disposizione dei nostri sindaci *(Commenti

esprimere due parole a nome del Gruppo Forza Italia su questo emendamento perché si tratta di uno di quei rari casi - o comunque non frequenti - in cui le forze politiche di maggioranza convergono con le forze politiche di opposizione realmente nell'interesse generale. Il tema Rigopiano, l'emendamento prevede di sostenere economicamente i bambini e le bambine resi orfani da quella tragedia che tutti quanti noi, credo, porteremo nel cuore e nella mente. È giusto che sia così perché uno Stato difficilmente può prevenire tragedie naturali come quella avvenuta a Rigopiano ma è dalla capacità, dalla qualità e dalla tempestività dell'intervento successivo che si misura la tempra di uno Stato e la qualità di chi ne ricopre le funzioni di Governo. È successo con Rigopiano, è successo, devo dire un po' malamente, con i genovesi colpiti dalla caduta del viadotto Morandi,

grave vizio, questa grave frattura all'interno del Parlamento, ma soprattutto all'interno del Paese, venga sanata. Vedo che il sottosegretario Crimi ha promosso un'indagine conoscitiva a otto mesi dall'insediamento del Governo, ed a oltre due anni e mezzo di distanza dai fatti. Confido quindi che prima o poi i partiti che sostengono questo Governo si chiariranno le idee su quello che è realmente necessario alle decine di migliaia di nostri connazionali colpiti, oltre due anni e mezzo fa, dal terremoto e che ci sarà prima o poi l'occasione per condividere degli emendamenti. Forza Italia ne ha presentati tanti: li abbiamo presentati in occasione del decreto terremoto, li abbiamo presentati in occasione del milleproroghe, li abbiamo ripresentati in occasione della legge di bilancio, e sono stati sempre respinti. Sono sicuro che arriverà il momento in cui verranno accolti e in cui potremo celebrare tutti insieme il senso dello Stato che ci dovrebbe appartenere.

siano le uniche figure importanti e determinanti del Servizio sanitario nazionale, ma perché in questo momento si stanno definendo i contratti. Qui c'è la possibilità di correggere un meccanismo che è nato da qualche anno, perverso e paradossale e forse nemmeno voluto dal legislatore che l'ha introdotto con il decreto Madia. progressivamente alcune quote già nel Fondo sanitario nazionale e già destinate agli stipendi dei medici vengono sottratte progressivamente negli anni, con un meccanismo complesso che chiaramente non riesco a spiegare qui. qui. Se questa erosione continuerà nel tempo, sarebbe inutile da parte nostra

sia in grado di mantenere le incentivazioni a restare nel Servizio sanitario nazionale, dobbiamo porre fine a questo meccanismo e a ciò è finalizzato l'emendamento in

relativo al cosiddetto emendamento trivelle, diventato noto - più o meno tristemente, a seconda dei punti di vista - negli ultimi giorni. Si tratta del vero motivo per cui il provvedimento in esame ha avuto un *iter* tanto travagliato, con imbarazzanti e imbarazzate continue richieste di rinvio. Bisognava che le due forze di maggioranza trovassero un accordo sulla materia: l'hanno trovato, ne hanno discusso a lungo, avranno anche un po' litigato e - come capita spesso in questi casi - hanno fatto un accordo al ribasso, un compromesso di bassissimo profilo, un *bluff* clamoroso, che adesso provano a vendere come un grande risultato. Invece non è nulla, se non un totale e insignificante accordicchio. che in Basilicata i 5 Stelle hanno fatto la campagna elettorale dicendo che, appena arrivati al Governo, sarebbero stati in grado di bloccare le trivellazioni e le coltivazioni di idrocarburi nella Val d'Agri: è assolutamente falso. L'emendamento che

Il ministro Di Maio aveva promesso di innalzare le *royalty* che vanno alle Regioni e ai territori locali e invece no: aumentano i canoni concessori, che vanno esclusivamente allo Stato centrale, per fare cassa, per i motivi noti, che conosciamo. Attenti, però, perché questa cassa è assolutamente incerta e rischia anzi di diventare un buco nel bilancio dello Stato, a causa dei contenziosi che si svilupperanno.

In compenso, mettete a rischio un settore, quello della ricerca scientifica, ingegneristica e tecnologia sull'*oil and gas*, in cui l'Italia è all'avanguardia, con posti di lavoro a repentaglio, come ha ricordato a tutti noi in questi giorni il sindaco di Ravenna. Non basta: cancellate la pubblica utilità, negando in tal modo un sacrosanto principio, ossia che la politica energetica sia eminentemente tema di carattere nazionale, che non può essere affidato ai territori locali. C'è di più, però: la politica energetica è un tema troppo serio perché possa essere affrontato nell'emendamento a un decreto-legge così ampio; anche a tale riguardo esprimo esprimo meraviglia, perché è stato ritenuto proponibile, mentre tanti altri sono stati cancellati. La politica energetica non può essere affidata a uno *spot* elettorale né a un emendamento *bluff*

guarderemo gli errori che continuate a fare.

quindi, l'azione che era necessario fare era evidentemente tutt'altra, come ci siamo permessi di dimostrare attraverso la presentazione di emendamenti e di subemendamenti che di fatto riscrivono completamente

per quanto riguarda la ricerca e la prospezione, e non con un inserimento all'ultimo minuto del famoso 4*-bis* - adesso è diventato comma 5 - anche delle istanze di concessione di coltivazione.

invece continuano ad andare avanti. Cito l'istanza di riattribuzione di concessione di coltivazione: Strangolagalli (Lazio, Frosinone); tre concessioni di 41,7 chilometri quadrati, e - se volete - vi dico anche chi ha presentato l'istanza. Cito l'istanza di concessione di coltivazione in Sicilia:

Facendo salve tutte le concessioni in essere - poi la chiamate moratoria -rimangono in piedi 116 concessioni di coltivazione in essere in Italia, che operano su un totale di 8.000 chilometri chilometri quadrati, tra cui: Basilicata, Puglia, Emilia-Romagna, Marche e Lombardia. Sono 66 le concessioni operanti sul fondale marino, su un totale di 8.064 chilometri quadrati.

di un piccolo passo in avanti, ma voi non potete assolutamente continuare a prendere in giro le persone e mistificare la realtà, perché questa non è una moratoria. Interviene solo parzialmente su alcune sospensioni. Voi pagherete dei prezzi per questo, perché non potete pensare di continuare a portare in giro gli elettori senza pagare pegno.

tradendo totalmente quello che avete detto e fatto in tutti gli anni precedenti.

Presidente, non voglio entrare nel merito specifico della questione, in quanto le sensibilità sull'argomento sono

La questione non è banale, perché - con tutto il rispetto per l'ambiente e il tema delle trivellazioni - sul piano politico, che regge le sorti di questo Governo, la questione è altrettanto importante.

parte, emendamenti vengono ritirati da uno dei *partner* di Governo - la Lega - e, dall'altra, vengono approvati quelli dell'altro *partner* di Governo, il MoVimento 5 Stelle.

speriamo che chi sta con voi metta cervello. Signor Presidente, sono intervenuto lungamente in discussione generale su questo tema, ma qualche risposta voglio dare a chi è intervenuto, ultimo ma non ultimo il senatore Mallegni. La capacità di mediazione politica e il compromesso parlamentare che si sono visti con questo emendamento dimostrano che questo Governo vi terrà all'opposizione per cinque anni. Questa è la prima La senatrice De Petris sa benissimo che No Triv, totalmente No Triv, in questa Aula siamo il MoVimento 5 Stelle e lei.

Mi va di dire qualcosa anche al senatore Margiotta, che chiama accordicchio un qualcosa che sospende la bellezza di 124 titoli

pagamenti, che peraltro possiamo ancora alzare, senza mai far pagare i cittadini, come ho detto ieri in discussione generale. Ma è anche una questione di giustizia sociale, Siete stati capaci di lasciare 5 milioni di poveri in Italia, ma mai vi siete permessi di toccare i petrolieri. Noi sì! Noi sì! Noi sì!

Dico che, sotto questo aspetto, abbiamo ottenuto un risultato enorme, secondo me. Oggi il PD dimostra ancora una volta quello che è e, come l'ultimo dei vigliacchi, non partecipa al voto.

Ho detto che si deve contenere. Non è ancora prevista la frusta, ma ci possiamo arrivare. La prego di non usare quelle parole, senatore

Se non lo capisce lei che ci lavora da tante settimane, figurarsi gli altri!

emendamento è stato votato prima, chiedo di rimetterlo in votazione e di fare una verifica.

rimane agli atti. Data la stanchezza di tutti e anche di chi è arrivato soltanto in questo momento, cerchiamo di procedere con tempi veloci ma utili per poter comprendere il prosieguo dei lavori.

sede confondere le istanze e cioè le richieste, con i procedimenti autorizzati non è bello: uno può presentare un'istanza e ritirarla; può presentarne a mazzi e ritirarle. Faccio, invece, notare al collega Castaldi che - per esempio - vengono fatti salvi tutti i procedimenti già in corso, anche se non si capisce a che livello del procedimento autorizzativo. Voi scrivete che «non si applica ai procedimenti in corso di conferimento di concessione». Ma che cosa vuol dire? dire? Quello di autorizzazione unica è un procedimento composito, fatto da procedimenti esterni ed endoprocedimenti; a quale punto non si applica? Dopo la prima conferenza di servizi? Dopo la richiesta di integrazione della conferenza? Al deposito del progetto definitivo? Prima della stesura del disciplinare di concessione? Dopo la consegna del disciplinare? Cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Senatore Coltorti, secondo lei, questo provvedimento...

che almeno su alcune questioni come l'*air gun* si potesse arrivare a un miglioramento. Torno a ripetere che questa non è una moratoria.

Prima di oggi, per quanto riguarda il mio impegno politico e giuridico, posso rivendicare il lavoro di una parte importante della Conferenza delle Regioni e in particolare delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia, quelle che hanno avuto un rapporto più stretto con il mare blu, con il mare Adriatico, che a più riprese ha conosciuto la pesantezza di questa difficoltà. Parlo con un *curriculum* di iniziative: siamo stati noi che abbiamo attivato *illo tempore* l'iniziativa referendaria, siamo stati noi che abbiamo attivato anche una interlocuzione con Palazzo Chigi a dicembre del 2015 per trovare una soluzione alla questione di Ombrina di ferro, che determinò una grande mobilitazione di persone, di giovani e financo di bambini. Arrivò in Abruzzo anche Erri De Luca a precisare la posizione che occorreva. Come si concilia questa norma, di cui adesso ci occupiamo pronunciandoci, con quello che serve per la difesa del mare blu? È una norma efficace? È una norma matura? è una norma frutto di un angolo, di un dialogo difficoltoso tra le due forze principali di Governo? È una norma che raccapezza, rimedia qualche centimetro di posizione politica e pubblica, che però non ce la fa a determinare la soluzione che è attesa dai Comuni bagnati dall'Adriatico, da coloro i quali vogliono un'altra maniera di approvvigionamento energetico. Io rivendico il lavoro fatto a dicembre del 2015 che portò alla morte di Ombrina di ferro. Concludo, Presidente, con una precisazione (non ho mai superato il tempo consentitomi): vorrei avere due voti, come disse una volta Ugo La Malfa, un voto per determinare l'allontanamento mio da una norma che non è efficace e un voto per incoraggiare una norma migliore, adulta, capace di fronteggiare il bisogno che abbiamo di mare blu, da una parte, e di approvvigionamento energetico, dall'altra. Per queste ragioni mi auguro che le Commissioni competenti, prevalentemente, si possono trovare fuori da ogni emergenza elettorale e da ogni esigenza di spettacolo tematico, per trovare una sede per dire una cosa

emendamento, perché non condividiamo né il metodo né il merito. Non condividiamo il metodo, perché non si può inserire in un decreto semplificazioni una norma di così grande impatto sociale e anche energetico e non condividiamo il merito, perché questo emendamento è praticamente la mediazione fra gli interessi politici della Lega e dei 5 Stelle che questa volta, mi perdonerà il collega Mallegni, vede il sopravvento della Lega rispetto al MoVimento 5 Stelle. Infatti, il collega Castaldi parla della sospensione di 120 autorizzazioni, ma lo invito a leggere il comma 5, in cui si dice che la sospensione di cui al comma 4 non opera nei confronti dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quindi fino a quando questa legge non sarà pubblicata ci potranno essere richieste di autorizzazioni che non potranno essere fermate.

Nel 2017 è stata approvata una strategia nazionale dell'energia di questo Paese. È legittimo che chi governa oggi possa voler modificare quella strategia, ma credo che di lì bisogna partire per poi arrivare alle ricadute sui singoli filoni e sui singoli settori. Noi oggi interveniamo prima delle trivelle, adesso sull'idroelettrico. Siamo intervenuti su altre forme di energia precedentemente, in modo puntuale, senza un disegno generale. Crediamo che questa sia una modalità, dal nostro punto di vista, non condivisibile. Sul tema puntuale di cui stiamo trattando, in senso generale, eravamo d'accordo: abbiamo presentato sia nella passata legislatura che in questa legislatura proposte normative che andavano esattamente in questa direzione.

modalità assolutamente non condivisibile, sbagliata nel metodo e nel merito, per cui non parteciperemo al voto di questo emendamento. Crediamo che sarebbe stato molto meglio quantomeno inserire questo testo nel testo base del decreto semplificazioni, in modo da permettere un minimo di confronto. Non c'è stato questo spazio, non c'è stato neanche lo spazio per fare un intervento decente in questa occasione.

di un'omissione del testo oppure questa intesa non è mai stata raggiunta? Se l'ipotesi fosse che questa intesa non è mai stata raggiunta, si tratterebbe di una norma che parte male, perché è una competenza concorrente, rispetto alla quale lo Stato non ha nessuna potestà legislativa piena, se non dopo aver avuto un confronto, nelle sedi istituzionali proprie, con le Regioni.

le strutture ricettive alberghiere, che hanno le stesse caratteristiche igienico-sanitarie, non possono somministrare alimenti e bevande alle persone che vengono da fuori o addirittura gli ospiti degli alloggiati. Questo è un Paese che guarda all'indietro, anziché guardare in avanti e questa è una misura contro il futuro e contro lo sviluppo, in un periodo di grande difficoltà e di crisi. L'emendamento propone una piccola cosa, per aiutare una delle più importanti imprese del nostro Paese, che è così meraviglioso.

La relatrice ha detto che è stato riformulato: ho cercato il testo preciso della riformulazione, perché vorrei capire intanto se nella riformazione rimane

in quanto i Comuni utilizzavano quel Fondo per la spesa corrente e invece, con la manovra di bilancio, viene destinato per opere di manutenzione, strade, scuole e strutture di proprietà comunale.

avranno la disponibilità di queste somme sul proprio bilancio dal giorno successivo all'approvazione della legge di conversione da parte delle Camere. È un risultato significativo che noi di Forza Italia vogliamo ascrivere a un lavoro importante e ringraziamo la

Apprezziamo il fatto che il Governo e la maggioranza abbiano deciso di procedere in senso totalmente diverso rispetto a quanto fatto nella legge di bilancio, che era piena di misure contro i Comuni. Nel frattempo è emersa la consapevolezza del danno arrecato e la volontà di porvi rimedio. Secondo noi, lo si fa in maniera insufficiente e in molti casi pasticciata, con troppi scaricabarile e incertezze, senza valorizzare pienamente il ruolo dei Comuni come propulsori della spesa per investimenti in Italia. La spesa per investimenti pubblici è sempre più determinante in un contesto di economia calante e occupazione in diminuzione. Tuttavia, la marcia indietro rispetto alla legge di bilancio ci è sufficiente per apprezzare lo sforzo fatto per correggersi e quindi ci asterremo.

su tutte le imprese del terzo settore, cioè su quella forza motrice del Paese che costituisce davvero l'asse portante del *welfare* italiano, un *welfare* creativo, delle opportunità e delle emergenze. Tassare in doppio modo quel tipo di attività era veramente la follia di un sistema che non si rendeva conto del valore delle iniziative. Da questo punto di vista, l'abolizione di questa tassa rappresenta un punto di civiltà nel nostro Paese.

Presidente, come con la legge di bilancio, ancora una volta maggioranza e Governo hanno mostrato incertezza e approssimazione nella conduzione dei lavori parlamentari. Nel caso di questo provvedimento, ciò è grave. Se infatti con la legge di bilancio c'era la trattativa con l'Europa, qui non c'è nulla che può spiegare quanto accaduto, se non le divisioni e i problemi tutti interni alla maggioranza, che non è riuscita a fare una sintesi virtuosa, senza cioè snaturare la funzione della decretazione d'urgenza. Per giorni e giorni la dialettica preminente è stata quella tra i due partiti di maggioranza e non quella tra maggioranza e opposizione. In attesa che altrove si prendessero decisioni e che venissero sciolti i nodi politici nelle Commissioni, abbiamo vissuto un *déjà vu* della manovra, come se nel frattempo non vi fossero state le parole di Mattarella, con il discorso di fine anno e l'invito alle forze politiche a riflettere sul ruolo del Parlamento. Il risultato di tutto questo è un testo finale fortemente al di sotto delle attese e delle necessità di cittadini e imprese. Come autonomisti avevamo presentato diverse proposte di buonsenso, condivise con le categorie produttive, che speriamo trovino spazio nella legge di iniziativa parlamentare che il Governo ha annunciato sulla materia degli appalti. Tra queste, quelle sulla modifica della disciplina del subappalto, con la soppressione della terna dei subappaltatori per ciascun servizio, l'introduzione di un termine di cinque giorni per la pubblicazione degli atti relativi alla procedura d'appalto, una revisione della norma sull'impugnazione dei provvedimenti per disincentivare i ricorsi di natura strumentale, un emendamento volto a scoraggiare le offerte con ribassi eccessivi e le offerte così basse da prefigurarsi come anomale, una proposta sul *rating* di impresa con la soppressione del soccorso istruttorio come criterio reputazionale. Sono solo alcuni esempi, ma voglio menzionarli, perché danno l'idea dell'importanza di un intervento su questa disciplina; spero davvero che, con il provvedimento *ad hoc* annunciato dal Governo, verrà concessa alle opposizioni una possibilità reale di confronto e di contributo. Il decreto-legge a nostro avviso ha comunque qualche aspetto positivo. Penso soprattutto alla cancellazione del Sistri, ma penso anche alla cosiddetta norma Bramini a tutela dei piccoli imprenditori che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Bene anche l'approvazione dell'emendamento, fortemente sostenuto dal nostro Gruppo, che ha riportato l'Ires per il volontariato al 12 per cento, riparando così al brutto errore compiuto con la legge di bilancio. Per il resto, non comprendiamo perché non sia stata accolta la richiesta, che giungeva da più parti, di superamento dello *split payment*. Era un intervento semplice, che avrebbe garantito maggiore liquidità alle imprese e ai professionisti, dato che oggi lo strumento cardine per il contrasto dell'evasione fiscale è la fatturazione elettronica. Quindi non capiamo perché il Governo non abbia voluto fare propria questa proposta. Ci colpisce che non abbia voluto confrontarsi sulla nostra proposta di semplificazione burocratica per la cancellazione automatica delle ipoteche, una volta saldati tutti i debiti. In questo caso sarebbe stata una norma a basso impatto per l'erario, ma aveva un suo valore simbolico, perché non è giusto che per un certificato che attesti ad esempio l'estinzione di un mutuo, i cittadini debbano pagare un'imposta di bollo di 59 euro. Ci colpisce ancora di più la bocciatura del nostro emendamento per estendere la disciplina dei *voucher* agli eventi sportivi internazionali, una richiesta che giungeva dal nostro territorio in vista dei campionati del mondo di biathlon del prossimo anno. Il punto è che per le società sportive professionistiche questa possibilità è consentita. Perché allora non estenderla anche alle associazioni e a quei soggetti *non profit* che organizzano eventi di così grande importanza? Parliamo di manifestazioni che smuovono migliaia di persone. Quest'anno, alla coppa del mondo, erano presenti oltre 100.000 persone in tre giorni. Sono eventi che generano ricchezza e sono straordinari veicoli di promozione del territorio e dell'Italia. Fa specie che la sua bocciatura sia giunta in concomitanza con la visita del Presidente del CONI a Bolzano, che ha definito la località Anterselva «asso nella manica» per la candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026. Allora, se non è una beffa la bocciatura di quest'emendamento, poco ci manca. Anche il settore dell'edilizia non ha trovato l'attenzione che merita, dalla mancata cancellazione dello *split payment* all'assenza di misure per l'edilizia infrastrutturale e le opere pubbliche. Mi sento allora di condividere quanto hanno detto i rappresentanti delle categorie produttive: questo provvedimento ha qualche elemento positivo, ma manca di un disegno sulla crescita e sullo sviluppo, la stessa mancanza che noi abbiamo sottolineato con la legge di bilancio. Le stime sulla crescita del Paese sono un terzo rispetto a quanto questo Governo scriveva nel DEF. Manca una vocazione all'impresa, allo sviluppo economico, che invece, in questo momento, dovrebbe essere molto forte, molto più decisa, molto più incisiva. Credo che un maggiore confronto parlamentare tra maggioranza e opposizione avrebbe aiutato in tal senso e ad evitare quello che è accaduto in queste ultime ore. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie.

l'*iter* della conversione di questo decreto-legge è stato, come sempre ormai, molto complesso; è stato, come al solito, pieno di problemi.

si era trasformato - già lo era in partenza - in una sorta di decreto *omnibus*. Come in tutti i decreti *omnibus*, ovviamente vi sono delle norme magari più positive ed altre, che sono state inserite e che avrebbero forse avuto bisogno di

Noi abbiamo cercato, in tutti questi lunghissimi giorni e settimane, di dare il nostro contributo. Abbiamo presentato emendamenti che entravano soprattutto nel merito di alcune questioni che

Speriamo, come abbiamo detto nell'intervento in dichiarazione di voto, che non ci si torni su, magari inventando qualche altra formula per colpire il volontariato. Spero che il voto di oggi fissi

e unicamente alle istanze per la ricerca e per la prospezione. Non vi rileggo l'elenco sterminato, ma si prorogano, ad esempio, tutte le concessioni in atto in Basilicata.

molte altre questioni che sono state poste in questa sede. Pensate al tema dell'idroelettrico: quella è una pubblicizzazione? È semplicemente un emendamento che favorisce ancora una volta la Lombardia (poi discuteremo su cosa accadrà con l'autonomia) e

Presidente, la semplificazione è un obiettivo primario per Fratelli d'Italia; la semplificazione arma le nostre azioni, investe il nostro impegno politico, è quello che ci viene chiesto dalla nostra gente, dalle nostre piccole medie aziende, dai nostri imprenditori, da chiunque voglia investire in questo Paese, questo Paese, dalla signora anziana che nei nostri paesi ci chiede aiuto perché nel 2019 il mostro è ancora la burocrazia.

In Commissione abbiamo dato la nostra massima disponibilità, ben presto tradita dalla vostra stella polare, che è così diversa dalla nostra. Voi avete dimostrato di avere come stella polare le elezioni europee, qualche comunicato roboante, qualche marchetta elettorale da lanciare sui *social.* Invece la nostra stella polare è l'interesse nazionale, è qualcosa di completamente diverso. Noi sappiamo quanto sia vitale semplificare e rendere più facile la vita dei cittadini e delle nostre imprese per poterle salvare dalle prescrizioni burocratiche e amministrative. Per questo abbiamo tentato di emendare, abbiamo tentato di dare una mano, abbiamo chiesto l'abolizione della fattura elettronica - vengo al sodo -, abbiamo chiesto l'abolizione del tetto del contante, che in Germania non esiste e in Italia continuiamo ad avere; abbiamo chiesto l'abolizione dello spesometro e del redditometro; abbiamo chiesto il reinserimento dei *voucher* per l'agricoltura e per il turismo; abbiamo chiesto la compensazione per chi ha crediti nei confronti della pubblica amministrazione, le tante aziende schiacciate, strozzate dai crediti che lo Stato non gli riconosce; abbiamo chiesto l'estensione del credito d'imposta previsto per alcune zone economiche, per il Sud,

pur occupandosi, come dicevo prima, di qualcosa per cui servirebbe un'enciclopedia per quanti volumi abbiamo dovuto trattare con tanta pazienza nelle Commissioni. Abbiamo parlato del codice degli appalti, del demanio delle acque interne, di scuola, di agricoltura, di ordini forensi, delle trivelle, per le quali ci siamo incredibilmente Abbiamo parlato della pubblica amministrazione, delle PMI, della tracciabilità dei rifiuti, dei medici, dell'Alitalia, degli enti locali, dei veterinari, dei concorsi pubblici. Fatemi dire due parole sull'Alitalia: vi sembra questo il modo di affrontare una questione come questa? Senza farci capire se esista la pianificazione di una strategia nazionale del trasporto aereo, del nostro sistema aeroportuale? Abbiamo visto - mentre qualcuno ride - stralciare fino all'ultimo istante due terzi degli emendamenti da noi presentati.

il tentativo positivo di mettere ordine nel caos delle licenze degli NCC e dei balneari. Abbiamo apprezzato gli aiuti a Rigopiano la norma sull'etichettatura con la quale si indica finalmente l'origine dei prodotti. Il resto è propaganda elettorale. Avremmo voluto votare a favore ma manca un ingrediente che per Fratelli d'Italia è fondamentale: il coraggio. Per questo il Gruppo Fratelli d'Italia si astiene su questo provvedimento. al nostro esame arriva in Aula in ritardo, com'è noto, dopo che l'Aula è stata bloccata per più settimane. Un decreto trasformato in *omnibus*, a serio rischio di costituzionalità, come abbiamo visto, rischio evitato *in extremis* dalle improponibilità e inammissibilità comunicate dalla Presidenza del Senato. La verità è che è in atto una campagna elettorale strisciante, una competizione tra forze di maggioranza sempre più antitetiche. Siamo stati bloccati a lungo mentre si cercavano mediazioni sempre più al ribasso. Il decreto-legge ha un titolo di sicuro effetto, in questo siete francamente bravi - dignità, sicurezza, spazza corrotti - ma dietro il titolo, anche in questo caso, nulla. Vi sfido anche questa volta a trovare che cosa possa giustificare il nome di semplificazione. Ieri è stato autorevolmente ricordato, in quest'Aula, l'articolo 77 della Costituzione ed il richiamo della Corte del 2012: nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme assolutamente ultronee rispetto al testo del decreto-legge. Ed invece il testo è cresciuto e lievitato di pari passo agli appetiti del Governo, intenzionato a far rientrare tutto quanto era stato tenuto fuori dalla legge di bilancio per le vicende della trattativa con Bruxelles a tutti note. Commissioni riunite sono state approvate 61 pagine di emendamenti, la stragrande maggioranza dei quali valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato, che questa volta ringrazio per la meticolosità del lavoro, credo anche supportata da autorevolissima *moral suasion.* Qui c'è un problema, che è quello di comunicazione tra i Presidenti delle Commissioni e la Presidenza del Senato: non possiamo per tre settimane votare emendamenti poi ritenuti inammissibili in Aula. Sono così scomparsi microinterventi, indegne mance, norme *ad personam*, provvidenze dovute a questo o a quel parlamentare per campagna elettorale. Qualche esempio? Un favore ad un operatore della logistica genovese, la modifica del CDA di ENAC per nominarne uno gradito al nuovo Presidente nominato solo dieci giorni fa, in coerenza con lo *spoil system* già esercitato su Ferrovie e su ANAS, di cui credo che il Governo sarà chiamato a rispondere dalla Corte dei conti; il potenziamento di Equitalia, non più ritenuto il diavolo come mesi fa, da quando l'amministratore delegato è di vostra nomina; persino un posto in più nell'organico del Ministero dell'interno; la pericolosissima deroga di tre anni concessa per l'adeguamento alla norma di sicurezza degli impianti antincendio nelle scuole, dove vivono i nostri figli, i bambini; l'incentivo alle un tempo odiate auto blu; la cancellazione del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e persino l'agghiacciante favore alle concessionarie, tra cui quelle autostradale e all'Aspi (a luglio bisognava togliere la concessione, oggi con un emendamento - poi per fortuna dichiarato inammissibile - in Commissione era stata approvata la deroga per le autostrade, tra cui l'Aspi, all'applicazione del codice degli appalti, evitando così il fastidio per loro di assegnare i lavori attraverso la gara). Altro che decreto semplificazioni: decreto complicazione, con molte norme ispirate solo da desiderio di potere, da voglia di occupare, con operazioni di sfacciato clientelismo, ogni spazio possibile. Un vero e proprio assalto alla diligenza. Ma qualcosa di buono c'è ed è grazie al PD - lo ha ricordato questa mattina il presidente Marcucci - ed è la cancellazione dello sbagliatissimo raddoppio dell'Ires sul *no profit*, un errore vostro nella legge di bilancio subito nominato «tassa sulla bontà». Vi diamo atto, su questo, di aver votato insieme a noi in Commissione prima e in Aula poi, un buon segnale, purtroppo episodico ed isolato, di corretta dinamica maggioranza-opposizione nell'interesse dei cittadini. Abbiamo convenuto insieme di evitare correzioni *spot* al codice degli appalti, una buona legge che certamente merita *check-up* e correzioni - sono il primo a dirlo - ma non certo stravolgimenti. però bocciato il nostro emendamento volto a cancellare l'aumento della soglia al di sotto della quale è possibile affidare lavori senza gara, una norma inserita nottetempo nella legge di bilancio, di cui Cantone ha detto che favorirà la corruzione. Quanto ipocrite suonano le parole di Bonafede e il decreto spazza corrotti, quando poi invece esiste uno iato evidente tra le vostre affermazioni e le vostre azioni. degli NCC e non mi dilungherò. Vi eravate impegnati ad affrontare il tema con una legge *ad hoc*, l'avevate presentata alla Camera e poi, mentre faceva il suo *iter*, l'avete rovesciata integralmente in questo decreto. Per pagare un dividendo politico ai tassisti, in particolare romani, schierati con la Raggi in campagna elettorale, colpite un settore che non è fatto solo di Uber o di grandi società, ma da tanti lavoratori autonomi, piccoli imprenditori che hanno investito soldi per poter lavorare. Le trivelle, un *bluff* clamoroso: promettevate di bloccare estrazioni e non bloccate niente; avreste dovuto aumentare le *royalty* che vanno alle Regioni e avete aumentato i canoni sperando di far cassa per lo Stato centrale e rischiando invece un buco serio causato da contenziosi. Non basta, mettete anche in ginocchio un settore - quello della ricerca e dell'ingegneria dell'oil and gas, in cui l'Italia è all'avanguardia. La chiosa più giusta alla vostra azione di Governo è in questa bellissima frase di Alexis «Le loro ambizioni sono talmente concentrate nel mantenimento del potere che, solo al pensiero di lasciarlo, sono presi da una sorta di orrore che impone loro di sacrificare l'avvenire al presente ed il loro onore al ruolo». Questo siete, ma non ve lo consentiremo, perché amiamo il nostro Paese.

stata ad ascoltare gli interventi dei colleghi: interventi anche importanti, che in parte ho condiviso in parte no. Non entrerò comunque nel merito del provvedimento in esame, che è già stato ampiamente illustrato in tutte le sue parti dai relatori e dal Governo.

Ebbene, ho trovato una nuova riforma degli enti locali, proposta con il decreto legislativo n. 78 del 2015, convertito con la legge n. 125 del 2015. In effetti, passò con un voto di fiducia, tanto alla Camera quanto al Senato, e precisamente con un maxiemendamento che sostituì interamente il testo. che aveva come contenuto la riforma degli enti locali, diventò un vero e proprio decreto *omnibus*: si partì dalla riforma della pubblica amministrazione e si arrivò a toccare la sanità. È lì, infatti, in quella riforma degli enti locali, che il Governo, con il maxiemendamento e la questione di fiducia, attuò la cosiddetta *spending review* sanitaria,

di anni di vera disattenzione politica da parte di chi ci ha preceduti. Ci impegniamo a cercare di risolvere magari con provvedimenti diversi, più piccoli, semplificati, ma lo faremo.

seduta delle Commissioni riunite viene convocata anche per il 15 gennaio e per il mercoledì, sempre alle ore 16 e alle 9, ma il 15 gennaio, dopo un'altra successiva comunicazione

per lunedì 21 gennaio, quando, improvvisamente, c'è una posticipazione della seduta dalla mattina al pomeriggio. Lo stesso 21 gennaio, nel pomeriggio inoltrato viene posticipata un'altra volta la seduta alle 20,30. Quando, poi, viene convocata - lo stesso giorno - per il giorno successivo alle 9,15, alle 9,59 c'è una sconvocazione per le 14,30 e le 17,30, e successivamente il giorno dopo... Insomma, ho ancora quattro fogli, mi fermo qua.

la realtà. Il tutto mescolato da una confusione di tipo politico, che ha visto questa maggioranza - ed entro nel tema politico - litigare nelle Commissioni riunite quasi su tutto. La maggioranza ha presentato oltre 400 emendamenti per poi ritirarli quasi tutti, o meglio sicuramente una parte della maggioranza - l'ho detto prima in un intervento - la Lega, ritira tutti

dal Gruppo FI-BP)*. Ma come si fa a non portare avanti queste cose? Dove è la politica di centrodestra? L'ho detto prima. Ho fatto i complimenti al MoVimento 5 Stelle: «siete stati bravi, vi siete portati via tutto».

sono anni che sentiamo ripetere la stessa cantilena secondo la quale il nostro Paese rischia di morire di passaggi burocratici: imprese, lavoratori autonomi, commercianti, agricoltori, artigiani, tutto il mondo produttivo conosce fin troppo bene quel calvario fatto di permessi che non arrivano, adempimenti che si susseguono, certificati, bolli e moduli che si accumulano. Uno spreco di risorse temporali ed economiche che spesso finisce per svilire anche il più strenuo dei cittadini. La burocrazia è una pesante *roulotte* che l'Italia si tira dietro da decenni e che le imprese non riescono più ad avere dietro come una zavorra. In termini assoluti, questo rappresenta oltretutto, come dice l'Istat, un'odiosa tassa occulta del valore di 31 miliardi di euro all'anno. Lo sappiamo da tempo immemore; eppure nelle precedenti legislature non si è fatto praticamente nulla per alleggerire questo carico burocratico che grava sui cittadini. Tante chiacchiere e zero fatti; si è continuato ad aggiungere quando invece era necessario togliere. Il MoVimento 5 Stelle lo sostiene da sempre e, con questo decreto-legge, fa un primo concreto passo per rendere più facile la vita agli italiani, a cominciare da quel male cronico rappresentato da uno Stato che non paga le piccole e medie imprese. E così la memoria va a cinque anni fa. Ricordate? Un giovane Presidente del Consiglio che oggi siede in quest'Aula, nel 2014, appena arrivato a Palazzo Chigi, dichiarò che avrebbe saldato in soli sei mesi - sentite bene: sei mesi - tutti i debiti che le pubbliche amministrazioni avevano con gli imprenditori. Ecco, Ecco, questa è stata solo la prima di un lungo filotto di promesse mai mantenute. Con questo provvedimento finalmente iniziamo ad invertire la rotta, con impegni concreti e non con le stanche promesse di Pulcinella, con cui la vecchia politica, quella dei supercompetenti che sanno tutto, ci ha riempito i timpani per anni. Oggi creiamo una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, finanziato inizialmente con 50 milioni di euro. Quando è certificato il legame tra la presenza di debiti che lo Stato ha nei confronti di un'impresa e l'impossibilità di quest'ultima di ripagare un prestito o un finanziamento, questa sezione speciale interviene a garanzia dell'imprenditore nei confronti della banca creditrice. Non si possono continuare a vedere aziende prigioniere del travaglio dei mancati pagamenti, con titolari di impresa che si tolgono il pane di bocca per tentare di sopravvivere. Proprio oggi uno studio ci dice che dal 2012 sono stati mille i suicidi per motivi economici nel nostro Paese. Ogni attività che chiude per la mancanza dello Stato è una sconfitta per tutti ed è giunta l'ora di fermare questa deriva. Il MoVimento 5 Stelle lavorerà notte e giorno in questa direzione. Pertanto, nel provvedimento che ci accingiamo ad approvare introduciamo nuove tutele a favore di chi fa impresa e si ritrova la casa pignorata per via della crisi. Accogliere il grido di dolore di Sergio Bramini era davvero il minimo che potevamo fare. Uno Stato che butta in mezzo a una strada i cittadini cui deve dei soldi non può e non potrà mai definirsi uno Stato civile. Due firme, quattro scartoffie, e ti toglievano via tutto: non si poteva più andare avanti così. D'ora in poi il giudice non potrà mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento delle somme dovute al cittadino; una novità di buon senso. Vogliamo un Paese che tuteli i suoi cittadini e che non diventi il loro aguzzino, come troppe volte è accaduto; le persone e la loro dignità devono venire prima di tutto. E veniamo al Sud. Da casertano ho smesso di contare i Ministri che negli anni si sono messi sulle labbra pirotecniche novità sul rilancio delle Regioni meridionali. Mentre il divario tra Nord e Sud aumentava di Governo in Governo, oltre al danno abbiamo dovuto sorbirci anche la beffa del fiume di parole inconcludenti della vecchia politica. In questo contesto sterile di annunci vuoti e di proclami altisonanti, sono nate, ormai da diversi anni, le zone economiche speciali in alcune Regioni del Mezzogiorno. Un proposito buono e lodevole, al quale però i "competenti" hanno abbinato una stupefacente siccità normativa, che ha reso del tutto stagnante il contesto economico delle aree beneficiarie di questa dicitura. Grazie al MoVimento 5 Stelle, tentiamo finalmente di far sì che le zone economiche speciali possano davvero cambiare marcia ed essere speciali di fatto e non soltanto di nome. Per le imprese che operano al loro interno vengono dimezzati i termini per il rilascio delle licenze, delle concessioni, dei permessi e di tanti altri passaggi burocratici. Inoltre, agevoliamo per esse anche gli interventi di urbanizzazione e istituiamo specifiche aree doganali in regime di sospensione IVA per le merci. Sono aiuti concreti, e non aria fritta venduta per svolta epocale, come si è visto troppe volte in passato; quella stessa aria fritta che ha attorniato per lunghi anni il percorso del Sistri. il Sistri, l'ardito e rivoluzionario sistemone che sempre loro, i sapientoni di turno competenti su tutto, ci avevano spacciato come panacea di tutti i mali per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Quello che è successo negli ultimi dieci anni è noto a tutti: un annuncio dietro l'altro, aziende del settore costrette a scucire moneta contante senza alcun ritorno, ed estenuanti e ripetuti rinvii. Un teatrino insopportabile rimasto in piedi per un decennio intorno a un meccanismo obsoleto, farraginoso e mai andato davvero a regime. Oggi chiudiamo questa inutile farsa politica. La tracciabilità dei rifiuti è un tema troppo serio per noi, e non lo si può derubricare a sberleffo normativo, come è stato fatto da troppi Governi. L'informatizzazione vera del ciclo dei rifiuti è una delle grandi sfide che ci attende nei prossimi anni: fermo restando un periodo transitorio, creeremo un registro elettronico nazionale presso il Ministero dell'ambiente, al quale le imprese dovranno iscriversi. Come tutti sapete, il MoVimento 5 Stelle è la forza politica che più di ogni altra crede nel progresso e nelle nuove opportunità che la tecnologia offre per migliorare la vita dei cittadini. Tra le tante novità che il decreto-legge prevede c'è l'ingresso della parola «*blockchain*» nel nostro ordinamento giuridico, che fa seguito ai 45 milioni di euro stanziati in manovra per dare il via a questa rivoluzione. E accanto al *blockchain* definiamo anche i primi contorni dello *smart contract*, un programma che opera su tecnologie basate su registri distribuiti come appunto il *blockchain*. È un'Italia che guarda avanti quella verso cui ci muoviamo con questo decreto-legge semplificazioni. E un'Italia che guarda avanti non può strizzare ancora l'occhio ai combustibili fossili.

Come il Movimento 5 Stelle sostiene da anni, è ora di dire sì alle energie rinnovabili, non solo a chiacchiere, ma in modo concreto, perché per ogni miliardo investito su fonti sostenibili possono nascere 13.000 nuovi posti di lavoro, a fronte delle poche migliaia che invece si creano trasformando in una groviera i nostri mari e territori trivellando a destra e a manca. Aspetto, questo, che demolisce ogni teoria economica di chi sostiene in modo miope e procelloso che con l'addio agli idrocarburi l'Italia rischia il baratro finanziario. Ovviamente non è così: sono soltanto gli ultimi sussulti di forze politiche e *lobby* petrolifere che spingono logiche energetiche ammuffite, pronte per essere consegnate ai faldoni della storia. Con questo provvedimento arrestiamo un gigantesco sfregio ambientale perpetrato per decenni in nome del profitto e ridiamo sovranità ai cittadini rispetto alle valli, alle coste, ai fondali, ai fiumi e a tutto ciò che fa dell'Italia il Paese più bello del mondo dal punto di vista naturalistico. Oggi aumentiamo di venticinque volte i canoni di concessione che le *major* petrolifere devono pagare allo Stato per svolgere le loro attività (oggi si pagano meno di 60 euro per coltivare idrocarburi per un anno su un chilometro quadrato di territorio). Soprattutto, sospendiamo tutti gli *iter* amministrativi per la concessione di permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi. Abbiamo fatto tutto questo discutendo in Commissione riga per riga, attraverso un'interlocuzione sana tra maggioranza e opposizione, che rappresenta l'*iter* con il quale, secondo noi, va licenziato un simile decreto-legge. Il MoVimento 5 Stelle, in ogni provvedimento che porta avanti in queste Aule, segue un'unica stella polare: quella che conduce al miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Per questo motivo, a nome di tutti i colleghi portavoce del MoVimento 5 Stelle, dico sì alle semplificazioni incluse in questo decreto-legge.